L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013». Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Enrico Signora Presidente, onorevoli senatori, è con profondo rammarico e profonda emozione che inizio questo intervento in quest'Aula sull'Europa, sul prossimo Consiglio europeo, ricordando ovviamente la figura di uno dei più grandi europeisti che l'Europa e il nostro Paese abbiano avuto, cioè l'ultimo Presidente italiano del Parlamento europeo: il vostro collega, senatore Emilio Colombo.

Solo poco più di quarantotto ore ci dividono ormai dal Consiglio europeo del 27 e 28 giugno. Negli ultimi cinquanta giorni ne abbiamo parlato a più riprese, in quest'Aula e nel dibattito pubblico. Lo abbiamo fatto sempre, sia pure con accenti e stili diversi, all'insegna di una consapevolezza condivisa: quello che ci attende sarà un duro confronto, un confronto importante, sarà un confronto tutto politico. Politiche vogliono e debbono essere dunque queste mie comunicazioni qui al Senato, così come politico sarà l'intervento di cui mi farò portatore dentro la sala del Consiglio europeo. Porrò l'accento, una volta ancora, sul dramma del lavoro che non c'è, sugli oltre 15 milioni di ragazzi senza un'occupazione, una prospettiva, un'opportunità di realizzazione, sull'Europa che o dà risposte concrete e immediate a problemi epocali come quelli che viviamo oppure lentamente muore. Un'Europa che stenta ad uscire dalla recessione, nella quale il livello degli investimenti pubblici è crollato negli ultimi anni e il rubinetto del credito bancario si è contratto drasticamente in alcuni Stati membri, tra cui l'Italia. Un'Europa che non riesce a riprendere velocità e nella quale le ombre sulla tenuta dell'Unione economica e monetaria non sono ancora state fugate del tutto. Sono bastate, in fondo, negli ultimi giorni, le notizie arrivate da Karlsruhe, sede della Corte costituzionale della

per riportare tensione sui mercati e far salire i tassi di interesse sul nostro debito. Sappiamo che il tempo stringe, quindi. Sappiamo che gli obiettivi fissati vanno realizzati al più presto. Sappiamo che dobbiamo contrastare la tendenza insidiosa all'inerzia, alla difesa ostinata di impostazioni rigide, alla protezione di prerogative nazionali e di egoismi nazionali. Sappiamo che, se si ferma, l'Europa, così com'è, è perduta. Da queste consapevolezze possiamo però ripartire nel prossimo Consiglio europeo. Al primo punto dell'agenda ci sarà, come sapete, la lotta alla disoccupazione giovanile. Ci si occuperà poi di finanziamento alle imprese e all'economia reale; ci si occuperà di riforme strutturali e di unione bancaria. Su tutti questi temi la risoluzione approvata dal Parlamento, da questo Parlamento, lo scorso 21 maggio, ha fatto da guida all'azione di preparazione e di negoziato che il Governo ha condotto nelle ultime settimane. Partiamo dunque dall'occupazione giovanile. È una realtà drammatica, la conosciamo benissimo: precariato, tutele disuguali, inattività. Su tutto, questo elevatissimo tasso di disoccupazione giovanile, che in Italia colpisce ormai il 40 per cento dei giovani tra i 15 e i 24 anni. È un dramma italiano, ma è un dramma anche europeo, collettivo, generazionale. Oggi in Europa un giovane su quattro è disoccupato. In alcuni Stati membri la soglia supera ormai il 50 un livello senza precedenti nel secondo dopoguerra. Per questo, fin dai primi momenti di vita del Governo, abbiamo fatto di tutto perché il tema diventasse centrale proprio nell'agenda del Consiglio europeo prossimo. È una scelta politica dirimente. Mi verrebbe da dire: è una scelta politica identitaria. Guardiamo per un istante indietro. Nella prima fase della crisi, in questi cinque anni, sono state compiute scelte che hanno mirato innanzitutto a proteggere, anche giustamente (le abbiamo fatte tutti insieme), il lavoro attuale e non certo quello futuro, il lavoro che c'era, il lavoro che si perdeva. Quella è stata la prima esigenza alla quale tutti insieme abbiamo fatto riferimento. Penso all'attenzione prioritaria che abbiamo attribuito alla tutela dei lavoratori già inseriti nel mercato del lavoro, con la cassa integrazione e gli ammortizzatori sociali. sociali. Contemporaneamente, penso alla riforma delle pensioni: anch'essa era necessaria, ovviamente, ma ha determinato un allungamento considerevole della vita professionale. Quindi, i giovani sono rimasti fuori, per l'una tendenza e per l'altra tendenza, non sono stati il centro dell'attenzione delle politiche del nostro *welfare*. Oggi non possiamo più ignorare questi squilibri. Non è solo la dimensione quantitativa della disoccupazione giovanile a preoccupare: è il rischio che diventi strutturale e letteralmente bruci un capitale umano prezioso e forse irripetibile. Eurofound ha stimato che il costo della disoccupazione giovanile in Europa, in termini di reddito perduto e di maggiori oneri di assistenza sociale, è pari a circa 153 miliardi di euro l'anno: una dissipazione senza pari. Come se non bastasse, vi è un prezzo meno visibile, ma più subdolo e grave da pagare. È il costo connesso alla creazione di una generazione tradita, e quindi ferita. Una generazione segnata da cicatrici profonde. Le cicatrici sulla comunità lasciate dalla frustrazione, dal risentimento e dalla rassegnazione sono le più difficili da cancellare, ed è su di esse che allignano e poi si propagano il populismo e l'antipolitica, l'ostilità verso le istituzioni pubbliche e verso l'Europa, la xenofobia, il rifiuto dell'integrazione. Per questo non potevamo accettare che il Consiglio europeo prossimo si fermasse a decisioni di *routine*, occupandosi soltanto di procedure, di *governance*, di tecnicismi, magari anche importanti, ma che non parlano al cuore dei cittadini europei, Ho voluto con tutte le forze che l'Italia non soltanto ponesse un problema politico, a nome del Parlamento italiano che questo mi aveva chiesto di fare, ma contribuisse anche con idee concrete. Abbiamo scritto al presidente del Consiglio europeo, Van Rompuy, il 24 maggio, inviando le proposte italiane per un'agenda europea di azioni contro la disoccupazione giovanile. Come sapete, almeno un primo traguardo è stato raggiunto: quello del lavoro giovanile, del lavoro per i giovani, adesso è un cardine della nuova agenda europea. È un risultato politico importante. Fare dell'occupazione giovanile un punto centrale di dibattito al Consiglio significa anche imprimere una direzione nuova alle scelte europee, in modo pragmatico, rifuggendo dal confronto semplicistico e inconcludente che spesso ha accompagnato la discussione europea. Volevamo lanciare un messaggio sull'anima sociale del vecchio Continente. Sei mesi fa si discuteva di finanze pubbliche, di tagli ai bilanci, di condizionalità per i programmi di assistenza degli Stati membri. Tutte questioni importanti. Oggi, però, ci si confronterà anche sulla formazione professionale, sugli investimenti sociali in capitale umano, sui finanziamenti alle imprese innovative create dai giovani. Il Governo italiano ha operato affinché in tutte le sedi europee maturasse la consapevolezza che promuovere l'occupazione per i giovani impone una maggiore integrazione tra politiche fiscali e politiche per il lavoro. È questo il senso dell'incontro che abbiamo organizzato e ospitato a Roma il 14 giugno scorso, presenti i Ministri delle finanze e del lavoro dei quattro più grandi Stati dell'area dell'euro: Francia, Germania, Spagna e Italia. È un formato che non ha precedenti nella dinamica europea: Ministri delle finanze e del lavoro insieme. Vuol dire che dalla centralità dell'Ecofin, in Europa bisogna passare sempre più alla centralità delle persone. Roma, per un giorno, è stata la capitale della lotta alla disoccupazione giovanile in Europa. Ora la capitale deve diventare itinerante: Bruxelles giovedì e venerdì e poi, il 3 luglio, Berlino, con un incontro dedicato anch'esso al lavoro per i giovani. L'Italia vuole essere in prima fila. Ne ha la volontà e ne ha anche la convenienza. Per questo domani il Consiglio dei ministri approverà alcune misure per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, aumentare l'occupazione, soprattutto quella giovanile, e sostenere le famiglie in difficoltà. Si tratta - voglio porlo in evidenza con grande chiarezza - di misure, quelle di domani, che saranno indipendenti da quanto avverrà nel Consiglio europeo: saranno scelte nostre, italiane, che sono evidentemente in sintonia con quanto si discuterà a Bruxelles. Forte di questa nostra iniziativa, chiederò con fermezza, che l'Unione non abbandoni a sé stessi gli Stati membri, ma ne supporti e rafforzi l'azione, mettendo in campo misure concrete, visibili ed effettive. Non è la prima volta che il Consiglio europeo affronta questi temi: lo ha fatto già nel marzo del 2005 con un Patto per la gioventù, che però poi ha avuto scarso seguito; ha fatto a più riprese nei mesi passati con dichiarazioni di valore soprattutto politico. Ora, chiediamo decisioni immediate che restituiscano il senso dell'urgenza, strumenti operativi europei e nazionali, risorse soprattutto, *tempi brevi per gli interventi* per ottenere il massimo dell'impatto subito. Come possono tradursi questi impegni? In primo luogo, facendo a livello europeo, che il modello della garanzia per i giovani, la *Youth Guarantee*, approvato dal Consiglio europeo ad aprile e che prevede che entro quattro mesi ogni giovane laureato riceva una offerta di lavoro, di studio o di apprendistato di qualità in Europa, diventi il parametro di riferimento per tutti gli Stati membri. Questo schema ha funzionato bene in Austria e in Finlandia: attuarlo in Italia comporterà una rivoluzione del nostro sistema delle politiche di attivazione e di orientamento al lavoro. Si tratta di un cambiamento tanto più agevole ed efficace, se attuato entro un quadro europeo certo. Per questo, nei prossimi mesi, anche alla luce di quanto sarà deciso a Bruxelles, vareremo un secondo pacchetto di interventi, proprio per dare attuazione alla garanzia per i giovani e per migliorare i servizi all'impiego. L'Europa dovrà mobilitare tutte le risorse disponibili. Chiediamo dunque di accelerare al massimo l'avvio dell'iniziativa europea per l'occupazione giovanile, un fondo istituito a febbraio scorso per il periodo 2014-2020, in modo che i primi progetti possano essere già finanziati a partire concretamente dal 1o gennaio 2014. Chiederemo però che l'uso di questo fondo sia concentrato nei primi due anni, e non più spalmato su sette. Sei miliardi di euro della garanzia significano circa 1.360 euro a disposizione di ciascuno dei potenziali beneficiari tra i giovani inattivi. È qualcosa, ma ovviamente non basta: per questo chiediamo che dal 2016 vi sia un rifinanziamento e un rafforzamento di questa misura per gli anni successivi. L'altra fonte di sostegno alle iniziative per i giovani sono, come è noto, i fondi strutturali, da cui arriveranno circa 55 miliardi di euro all'Italia nei prossimi sette anni. Chiediamo che nella nuova programmazione la promozione di lavoro per i giovani abbia la priorità, così come riteniamo importante l'utilizzo del Fondo sociale europeo per finanziare incentivi all'assunzione dei giovani, anche mediante la riduzione del cuneo fiscale, che per noi rimane la grande priorità. Vogliamo inoltre che l'Unione europea usi in modo mirato una delle sue carte migliori, finora poco e male utilizzata: la Banca europea per gli investimenti. Chiediamo che la BEI aumenti il credito erogato alle piccole e medie imprese, che rappresentano il cuore del nostro tessuto produttivo (attualmente questo vale circa 13 miliardi di euro). Bisogna sviluppare strumenti specifici volti a sostenere l'occupazione giovanile e gli investimenti pubblici nella formazione professionale e nell'istruzione, anche in coordinamento con le istituzioni finanziarie nazionali, come ad esempio la Cassa depositi e prestiti. chiediamo passi avanti in ordine alle misure per facilitare la mobilità geografica dei lavoratori: la mobilità europea dei giovani è nei fatti, ma ancora siamo lontani da un mercato unico del lavoro. le parti sociali possono apportare un contributo determinante. Ho avuto modo di incontrare i sindacati italiani ieri mattina, incontrerò i sindacati europei giovedì mattina a Bruxelles e

a livello europeo, che saranno presenti, interverranno, porranno la loro posizione. Questo sarà un fatto, secondo noi, sicuramente importante e innovativo rispetto a tutti questi temi. D'altra parte, con franchezza dobbiamo ribadire che, se l'Europa non riprende un cammino di crescita, nessuna delle decisioni puntuali che potremo assumere condurrà a una vera svolta. Su questo entra in gioco il secondo punto in agenda al Consiglio: la verifica dei progressi compiuti nell'attuazione del Patto per la crescita e per l'occupazione, adottato nel giugno 2012, principalmente su impulso del Governo presieduto da Mario Monti. A un anno esatto di distanza, il bilancio europeo di quelle scelte è a luci e a ombre. Nel campo del mercato unico sono stati compiuti progressi importanti, ma un buon numero di misure è ancora bloccato, benché il termine fissato a dicembre 2012 sia ormai scaduto da alcuni mesi. In altri settori, dall'energia all'area europea della ricerca, molto resta da fare. L'aspetto centrale del Patto è, tuttavia, l'accento posto sull'uso della Banca europea per gli investimenti come leva per fare ripartire gli investimenti produttivi. A tal fine, era stato deciso l'aumento di capitale della stessa BEI, che è stato completato positivamente nei primi mesi del 2013. A regime, l'aumento di capitale permetterà di aumentare i prestiti della BEI negli anni 2013-2015 di 60 miliardi, mobilitando così oltre 120 miliardi di nuovi investimenti in tutta Europa. Dal nostro punto di vista la discussione sulla politica di investimento della BEI costituirà, dunque, uno degli snodi del Consiglio europeo. Essa può avere un ruolo chiave nel catalizzare risorse per investimenti di lungo termine; soprattutto è il potenziale perno di un'azione volta a riattivare il credito per l'economia reale e a contrastare la frammentazione dei mercati finanziari. Del resto, oggi, in Europa, le condizioni del credito alle imprese divergono sensibilmente da Stato a Stato, perché riflettono non solo il merito di credito delle singole imprese, ma anche la loro posizione geografica. È una situazione che penalizza le imprese italiane e quelle di altri Stati membri. Ci batteremo, dunque, per un ruolo più deciso e incisivo della Banca europea per gli investimenti a sostegno dell'economia reale e delle piccole e medie imprese, che più hanno bisogno di credito per investimenti. Più in generale, i progressi sul fronte della crescita sono legati alla capacità di tenere la rotta delle riforme strutturali. Il Consiglio europeo affronterà come terzo punto l'esame delle raccomandazioni della Commissione europea ai Paesi membri, portando a conclusione il semestre europeo 2013. Non è un passaggio solo procedurale: il semestre europeo è positivo perché aiuta a coordinare le agende nazionali per le riforme. Dobbiamo contribuire a consolidare questo esercizio. Lo prendiamo, del resto, molto sul serio e, come più volte ho ribadito, interpretiamo le sei raccomandazioni che la Commissione ci ha rivolto - in parallelo con la positiva chiusura della procedura per *deficit* eccessivo - come la base della nostra azione di governo. A ben vedere, abbiamo già iniziato a farlo con i provvedimenti adottati nelle ultime settimane: penso alle norme per l'accelerazione della giustizia civile; penso al pacchetto di misure sulle infrastrutture; penso alle semplificazioni, agli interventi sul credito contenuti nel «decreto fare» e che incrociano puntualmente le raccomandazioni della Commissione. Allo stesso modo, il disegno di legge sulle semplificazioni e il decreto-legge sull'occupazione giovanile, che approveremo domani, rispondono a sollecitazioni che vengono anche dalla stessa Unione Dobbiamo poi procedere con maggiore attenzione e sistematicità all'attuazione delle direttive europee. Per questo sono lieto che il Senato abbia calendarizzato già per la prossima settimana l'esame in Aula della legge europea 2013, attualmente all'esame della Commissione politiche dell'Unione europea. Mi auguro che si possa chiudere rapidamente l'*iter* di approvazione di questo disegno di legge, che contiene norme necessarie per il recepimento delle direttive dal 2011 al 2013, ed evitare il Governo, coordinato su questo tema dal ministro Moavero, sta facendo un gran lavoro - il massimo numero di procedure di infrazione. Vengo adesso all'unione bancaria, e più in generale alla riforma della *governance* dell'Unione economica e monetaria: il quarto punto sull'agenda del Consiglio. In questo campo, soprattutto sull'unione bancaria, il cammino è accidentato e ancora in salita; si stanno finalizzando, con fatica, i primi passi: dopo l'accordo sul meccanismo unico di supervisione bancaria e sulle linee guida per la ricapitalizzazione diretta delle banche da parte dell'*European Stability Mechanism* si cercherà di chiudere un accordo sulla direttiva in materia di risoluzione ordinata delle crisi bancarie e, a cascata, sulla direttiva relativa alla garanzia, a favore dei risparmiatori, dei depositi bancari. Su tali temi, l'Italia è impegnata a respingere le obiezioni di chi dà l'impressione di non voler veramente progredire, ma anche ad offrire soluzioni per mediare tra interessi difficili da comporre. Un dato è, comunque, certo: a Bruxelles, a nome del Governo italiano, ci batteremo perché non si rimetta in alcun modo in discussione il calendario deciso dal Consiglio europeo di dicembre per completare l'unione bancaria, faremo di tutto affinché vi sia al più presto una proposta della Commissione per un meccanismo comune di risoluzione delle crisi bancarie e si arrivi all'adozione entro l'attuale mandato del Parlamento europeo. Tutto ciò farà da base per la grande battaglia politica per l'Europa che inizieremo dall'autunno, in preparazione dell'occasione unica che all'Italia si presenterà nel 2014: il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea nella seconda metà del 2014 potrà rappresentare, come indica la risoluzione qui presentata, l'opportunità per porre le questioni istituzionali e la dimensione politica al centro dell'azione dell'Unione e degli Stati membri. L'occasione è unica per dare il via, proprio dall'Italia, alla costruzione degli Stati Uniti d'Europa, idealità alta e ineludibile per le attuali generazioni, sola bussola e solo orizzonte della politica europea di un Paese come il nostro. Infine, Consiglio europeo assumerà decisioni importanti in materia di allargamento. Saluteremo l'ingresso della Croazia come Stato membro dal 1° luglio;

Ci pronunceremo sulla proposta della Commissione di aprire i negoziati per l'adesione della Serbia, auspicando che sia fissata subito una data per l'avvio dei negoziati stessi. Croazia, Lettonia, Serbia: tre casi diversi di avvicinamento all'Europa all'Europa unita e a tutto ciò che essa storicamente rappresenta; tre esperienze per ricordarci che l'Unione europea era e resta una storia di successo. La crisi e i tanti, troppi, errori commessi nell'ultimo decennio tendono a farcelo dimenticare, ci inducono a focalizzare l'attenzione e i nostri umori su tutto ciò che non funziona: sull'austerità, sulle lentezze procedurali, sull'incapacità di decidere per il meglio. Ed è vero, certo, ma l'Europa non può essere soltanto questo. Solo insieme, dentro l'Unione, possiamo raggiungere risultati che altrimenti, da soli, non potremmo neanche progettare. Sul punto, permettetemi un aggancio alla recentissima esperienza vissuta al G8. Lì abbiamo verificato cosa può davvero fare l'Europa quando non è più sul banco degli imputati, ma voce unitaria al tavolo globale. Lì si è assunta la storica decisione di avviare i negoziati per un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti: è un accordo che può dischiudere prospettive economiche nuove, facendo crescere il PIL europeo dello 0,5 per cento l'anno, e che ha un significato geopolitico rilevante. rilevante. Secondo tutti gli studi, l'Italia è il Paese che ne avrà più vantaggi, proprio per il tipo di economia aperta che abbiamo. Ci auguriamo che tale accordo possa essere chiuso proprio sotto la Presidenza italiana. Signora Presidente, onorevoli senatori, ora sta a noi, rappresentanti del popolo italiano, qui, e delegati dai popoli europei, giovedì e venerdì a Bruxelles: possiamo e dobbiamo decidere per costruire qualcosa di più forte e solido, e non per tamponare un'emergenza. Cercheremo di cogliere questa opportunità, rifuggendo da ogni soluzione al ribasso. Il nostro impegno, il mio impegno, è quello di trasferire ai *partner* europei una sola urgenza: dare finalmente risposte vere, concrete, subito verificabili, ai problemi dell'Europa dei popoli, e il primo problema, oggi, è il lavoro che non c'è per milioni e milioni di ragazze e ragazzi. A loro abbiamo l'obbligo di indicare una rotta e di restituire, finalmente, una speranza.

Signora Presidente, mi consenta di iniziare associandomi alle parole del Presidente del Consiglio nel ricordo di un grande europeista, di un grande collega, che ha presieduto la prima seduta di questa legislatura, qui al Senato, ed anche al Senato, ed anche la Commissione esteri, ricordandoci il suo sogno: quello degli Stati Uniti d'Europa. Emilio Colombo è stato un grande protagonista della vita pubblica italiana ed europea, e credo che il nostro Parlamento avrà modo L'Italia ha fatto la sua parte: l'hanno fatta anzitutto i cittadini italiani con i sacrifici che si sono sobbarcati in questi mesi; l'ha fatta per merito anche del Governo Monti - mi sembra giusto ricordarlo, perché è stato un frutto comune tra le forze politiche

L'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo aperta nei nostri confronti nel gennaio del 2010 ci consente oggi di poter guardare con maggiori margini di manovra al nostro futuro. Nessuno di noi viene dalla luna e tutti dobbiamo essere consci delle responsabilità passate e delle sei raccomandazioni che la Commissione europea ci ha rivolto. Non basta, senatori, la riforma dell'articolo 81 della Costituzione. Bisogna insistere - lo ha detto il Presidente del Consiglio

che a questo punto una grande responsabilità in proposito l'abbia proprio il Ministro dell'economia, che qui salutiamo: il ministro Saccomanni. A questo punto, oggi, senza ripetere le tante cose illustrate dal Presidente del Consiglio su cui sono e siamo d'accordo, io penso che bisogna andare al nocciolo dei problemi. Qui, oggi, entra in ballo la responsabilità dell'Europa, che non può limitarsi solo a controllare in modo ragionieristico i nostri parametri imponendoci rigore. Come dimostra la nostra situazione (e non mi riferisco solo all'Italia), di solo rigore e austerità si può anche morire. Il presidente Letta ha parlato di un confronto che avrà a Bruxelles, e lo ha definito un confronto duro, un confronto su basi politiche. Io credo che sia proprio così. Il nostro Paese deve prepararsi a un confronto duro, a un confronto politico. L'esperienza americana ci deve indurre a riflessioni sistemiche. Non va fatta cadere, ad esempio, la proposta di valutare il rispetto del Patto di stabilità ogni tre anni, invece che ogni anno, facendo una media, perché in alcuni momenti il *deficit* può essere necessario. Peraltro, i dati dell'ISTAT dei primi tre mesi di quest'anno sull'*export* italiano ci dimostrano che si sta allargando la debolezza economica a tutta l'area dell'euro, compresa la Germania, flettono le nostre esportazioni, si allarga il contagio anche agli altri Paesi. Fino a ieri, forse, c'era l'illusione di qualche Paese europeo, in particolare della Germania, che la crisi potesse essere limitata ad alcuni Paesi alcuni Paesi dell'area mediterranea. I fatti purtroppo ci inducono a dire che non è così, che è una illusione nella quale si sono cullati gli stessi colleghi della Germania. Sottoscriviamo dalla A alla Z le proposte del Governo sull'occupazione, in particolare quella giovanile, ma non ci sarà la soluzione del problema senza la capacità di sciogliere altri nodi. Le richieste italiane di escludere una serie di investimenti strutturali dal calcolo del disavanzo non hanno ancora avuto le risposte che meritavano. Su questo si può fare di più, magari calcolando percentuali diverse sul prodotto interno L'unione bancaria ha fatto un passo avanti sul meccanismo di supervisione comune, ma anche un passo laterale sull'utilizzo del meccanismo di stabilità per ricapitalizzare le banche e un passo indietro sui meccanismi comuni per la soluzione delle crisi bancarie. La guida dell'Unione - lo dico con chiarezza assunta da un direttorio franco‑tedesco che sia fondato, come emerge nel recente documento comune, su un accordo avente come principale denominatore comune il rinvio delle riforme: il rinvio delle riforme strutturali interne in Francia contro il rinvio della riforma dell'unione bancaria, che suscita qualche perplessità in Germania. Si parla - e lo ha fatto il Presidente del Consiglio - di mercato unico del lavoro, si parla di mobilità. Purtroppo la mobilità è già ampiamente avviata, ma per ora riguarda soprattutto lavoratori con livelli di istruzione elevata. È quella che noi chiamiamo la fuga dei cervelli, che non ci stanchiamo di evocare come un elemento di debolezza del nostro sistema Paese.

Ha fatto bene il Presidente del Consiglio a dire, in diversi suoi interventi, che si deve trattare di mobilità circolare, che non deve essere una pura fuga di risorse umane per il nostro Paese. Finora per noi questa mobilità del lavoro ha significato soprattutto spostamento di lavoratori italiani, così come di lavoratori greci o di altri Paesi in difficoltà verso Paesi dell'Europa del Nord e in Germania. Resta il fatto proprio per le qualifiche più basse, proprio per i lavoratori meno specializzati, la mobilità dei lavoratori è un modo più elegante e politicamente corretto di chiamare l'emigrazione. Certo, è una emigrazione diversa dal passato, perché c'è la cittadinanza europea, c'è Internet, ci sono i voli *low cost*, ma sempre di emigrazione si tratta. Se l'unica strada per sconfiggere la disoccupazione è l'emigrazione, significa che siamo davvero con le spalle al muro. Infine, il Parlamento italiano si impegna - come è scritto nella risoluzione n. 5 di maggioranza, che ho sottoscritto - a promuovere la convocazione di assise sull'avvenire dell'Europa, una grande riunione parlamentare di rappresentanti di popolo che sia capace di dare uno stimolo di idee, proposte e impegno per la ricostruzione dell'Europa politica. Anche questa iniziativa di domani potrà essere coronata da successo se i Governi sapranno nelle prossime ore, ossia oggi, affrontare positivamente le questioni concrete sul tappeto, a partire dal delicato negoziato sul prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea. In caso contrario, colleghi, dico con chiarezza che non vorrei che trasformassimo l'assise auspicata in un ennesimo esibizionismo di euroretorica: l'euroretorica, oggi, è il vero ricostituente per i movimenti populisti antieuropei che si moltiplicano nel Continente. È un'impresa difficile, ed io credo che, a prescindere da ogni altra considerazione, l'appoggio convergente di forze politiche diverse, tra loro anche alternative, che si registra attorno al Governo, trovi la sua motivazione principale nell'asperità e nella difficoltà di questo momento. Non è un momento che l'Italia può affrontare da sola fuori dal quadro europeo. Se l'Europa non cambia passo, se non trova in questo momento la capacità di una condivisione di destino comune, nulla sarà possibile per il nostro Paese. Chi come me e come tanti altri in quest'Aula coltiva da sempre il sogno dell'europeismo non può affidarsi solo agli atti di fede. Gli atti di coraggio devono avere la capacità di poggiare su azioni concrete e significative. Penso che si debba augurare al Presidente del Consiglio in bocca al lupo, sapendo che in questo caso c'è dietro di lui tutta l'Italia*.

negli anni del Governo Prodi e poi in questi ultimi, frequenti rapporti ed ho apprezzato il suo senso delle istituzioni, la sua semplicità nei rapporti con le persone, il suo impegno sui grandi valori della nostra Costituzione.

i punti indicati, le proposte e le iniziative che il nostro Governo vuole portare avanti. Voglio soprattutto richiamare due temi: il primo è quello su cui il nostro Governo ha insistito e che è riuscito ad inserire con forza all'ordine del giorno di questo Consiglio europeo.

dobbiamo promuovere misure urgenti, fare un cambio di passo e una svolta. Una svolta naturalmente legata ad un rapporto stretto che deve esserci tra piano per il lavoro, piano per l'occupazione e piano per lo sviluppo. Infatti nessuna misura di sostegno all'occupazione, anche a quella giovanile, nessuna misura

Quindi, dobbiamo promuovere questa svolta. Sono d'accordo con quanto sottolineato ora dal presidente Casini: una cosa è la revisione della spesa pubblica, che dobbiamo realizzare, e una cosa sono il rigore e l'efficienza, che ci dobbiamo imporre, ma di sola austerità si muore. Se c'è soltanto l'austerità - come si vede - si colpiscono i ceti popolari, i ceti più deboli, la speranza dei giovani nel futuro. E se vi sarà una rottura definitiva tra speranza delle giovani generazioni e prospettiva dell'Unione europea come grande democrazia sovranazionale, tutti quanti arretreremo, e non di poco.

utilizziamo le risorse che abbiamo ‑ e non quelle che vorremmo ‑ finalizzandole a questi temi dà credibilità a questo impegno. Voglio concludere su questo punto ricordando, però, oltre a quelle che lei ha citato, altre due misure:

essere credibili e coerenti: dobbiamo fare in modo che siano premiati i Comuni e le Regioni che hanno avanzi di amministrazione. Se qualcuno di questi enti ha un avanzo di amministrazione e ne può spendere una parte per queste finalità, allora la virtù funziona, altrimenti diventa una notte indistinta

che caratterizzerà fortemente il semestre in cui noi guideremo il Consiglio europeo. Anche da parte mia, signor Presidente, in bocca al lupo per il Consiglio europeo.

anche il nostro Gruppo si inchina commosso alla memoria di Emilio Colombo, un grande italiano, un grande europeo, che ci ha lasciato, nelle fatiche del suo ultimo volume «Per l'Italia, per l'Europa», non soltanto una testimonianza, ma anche un libro carico di indicazioni, di cui mi auguro che quest'Aula possa al più presto far tesoro. Quanto alle comunicazioni che ha reso il Presidente del Consiglio, noi ci vediamo una speranza: la speranza che giovedì e venerdì suonino davvero in Europa le campane (addirittura, le fanfare) di un grande e irrinunciabile accordo per combattere la disoccupazione giovanile. Ma nel nostro animo c'è anche la preoccupazione registrare, giovedì e venerdì, l'ennesima perdita di sovranità nazionale senza che essa sia compensata da meccanismi comunitari o, come diceva il collega Chiti, intergovernativi più efficaci. Tra questa speranza e questa preoccupazione, c'è un po' lo stato d'animo con il quale il rapporto fra il nostro Paese e l'Europa, l'Europa e il nostro Paese si è andato atteggiando negli ultimi tempi. Quale fu, colleghi senatori, il vero limite del Trattato sul *fiscal compact* inerente la politica di bilancio degli Stati firmatari? E lasciamo perdere, se ci riusciamo, la disputa fra le opposte tifoserie su quante responsabilità abbia avuto il berluscon-tremontismo a firmarlo e il montismo a farcelo approvare. La verità è che con quel trattato aumentava considerevolmente il livello di disciplina sui bilanci nazionali e si riducevano i margini di discrezionalità dei Paesi della cosiddetta periferia europea. Casini evocava l'Europa mediterranea. Oggi esiste un'Europa molto sbilanciata fra un baricentro settentrionale e la condizione dei Paesi mediterranei.

a negoziare di continuo, ininterrottamente, concessioni (e lo dico fra virgolette) con le autorità europee. Metto queste virgolette perché l'Europa è una costruzione del secondo dopoguerra democratico; è una costruzione nella quale ci sono diritti che si ottengono, non diritti che si concedono, come nella restaurazione post-napoleonica del 1814. Da questo punto di vista, colleghi senatori, pensiamo al caso dei pagamenti arretrati dovuti dalla nostra pubblica amministrazione, che è stato in qualche momento un incubo del nostro rapporto con l'Europa. Da questo punto di vista non c'è dubbio che l'unione bancaria, ha fatto bene a registrare, ha compiuto passi avanti, passi indietro e passi di lato. O è una costruzione europea o, se deve essere soltanto una costruzione tutta e soltanto tedesca, se la tengano i tecnocrati, che nella storia dell'idea d'Europa possono avere un utile ruolo di fiancheggiamento, ma non possono pretendere di svuotare quel primato della politica che con De Gasperi, con Giscard d'Estaing, con Kohl, con lo stesso Mitterrand ha suonato alto e forte nei momenti migliori di questa costruzione. Onorevole Presidente del Consiglio, lei ha tratteggiato in modo molto articolato quali sono i punti attraverso i quali è auspicabile che il vertice europeo possa rilanciare crescita e occupazione. Del resto, già da qualche giorno la Commissione ha varato la riforma Almunia sugli aiuti agli investimenti delle imprese. Ne ho appreso qualcosa da un articolo di Adriana Cerretelli su «Il Sole 24 Ore» di domenica. La riforma Almunia traccia una sorta di nuova disciplina della distribuzione delle risorse fra i vari ordinamenti regionali. Quasi un nuovo codice - si parla di codice Almunia su «Il Sole 24 Ore» - che serve a ripianare il divario tra Nord e Sud dell'Unione europea. Ed è importante la determinazione, l'impegno e la serietà con la quale il commissario europeo all'industria Antonio Tajani ed altri 13 suoi colleghi,

a quella che il Presidente del Consiglio chiamava l'Europa sociale, mai contrapposta nella sua storia, e credo nel suo futuro, all'anima liberale dell'Europa. Non so quanto l'Italia possa giovarsi di questo codice Almunia. Vi era il rischio che venissero irrimediabilmente fermate le Regioni della fascia A. La Lombardia e il Veneto, colleghi della Lega. Ma noi siamo meridionali, meridionalisti, e abbiamo sempre considerato la nostra come una grande questione nazionale: non si tratta di fermare il Nord, il Nord, ma di far valere delle priorità meridionali. Stamattina mi è dispiaciuto vedere con quanta sciatteria alcuni colleghi hanno fatto riferimento

Politica istituzionale, se vuole politica costituzionale, e politica economica si legano negli obiettivi del suo Governo.

Un ordinamento regionale con 21 Regioni incapaci di spendere, non ce lo possiamo assolutamente permettere. C'è bisogno di forti correttivi costituzionali.

il torbido gioco dei localismi (Reggio Calabria contro Catanzaro, Pescara contro L'Aquila, Avellino e Benevento contro Napoli). Da questo punto di vista, onorevole Presidente del Consiglio, il nostro regionalismo doveva essere di legislazione e programmazione e non di gestione. Apprendiamo dall'ex ministro Moavero che questa gestione è pessima. È una preoccupazione che non ci rafforza nel nostro modo di stare e voler bene all'Europa. Signora Presidente, Presidente del Consiglio, Ministri, colleghi, con questo mio intervento vorrei richiamare la vostra attenzione su un aspetto specifico della relazione programmatica oggi in discussione, quella della fiscalità. Tuttavia, le mie considerazioni non saranno sul merito, ma sulla grammatica. Sul merito, infatti, non si può negare che il documento proposto contenga proposte e intenti in buona parte condivisibili, volti principalmente alla semplificazione e all'armonizzazione dei sistemi impositivi, nonché al contrasto dell'ormai endemico fenomeno dell'evasione fiscale. Si pone anche l'accento, forse per la prima volta in maniera netta a livello europeo, su un altro fenomeno, che nel nostro Paese è ben noto e che crea danni pari se non superiori all'evasione fiscale: l'elusione fiscale. D'altronde, come confermato anche in un recentissimo convegno dell'Associazione nazionale ufficiali di complemento e riservisti finanzieri, tenutosi proprio a Roma, il termine «elusione fiscale» in ambito europeo spesso risulta sconosciuto e viene sostituito con un più diplomatico *aggressive tax planning*, ovvero pianificazione fiscale aggressiva. Su questo tema, evidentemente - e aggiungerei purtroppo - il nostro Paese è all'avanguardia. altro elemento positivo, che emerge scorrendo le pagine della relazione, è costituito dalla sensibilità e dall'impegno propulsivo che l'Italia - Paese spesso guardato con sospetto e magari iscritto nelle liste dei cattivi in ambito internazionale - dimostra di avere su alcune delle tematiche in oggetto. Tuttavia, come ho detto, voglio soffermarmi sulla grammatica. Sin dalle prime pagine è impossibile non notare come questo documento sia il trionfo del condizionale - si trova scritto: «dovrebbe», «potrebbe» - e tra quelli utilizzati frequentemente appaiono i termini «veto», «riserva», «contrarietà».

signor presidente Letta, un passaggio della sua interlocuzione con il sottoscritto, relativa al suo intervento del maggio scorso, in questa Camera, in occasione del Consiglio europeo del 22 maggio. Riferendosi in particolare ai paradisi fiscali,

signor Presidente, chiedo a me stesso, a lei e a questa Assemblea: siamo sicuri che si tratti sempre di ipocrisia? Siamo sicuri che in questi Paesi, la cui economia innegabilmente è sempre stata trainante per l'economia dell'intero sistema Europa, non si sia alla fine sviluppata la consapevolezza che in questa Europa alcune regole vanno bene per qualcuno, ma non per tutti, e che quel qualcuno non è necessariamente uno dei Paesi in maggiore difficoltà? la consapevolezza che il processo di unificazione sia iniziato da quello che sarebbe dovuto essere l'ultimo passaggio e avrebbe dovuto seguire un'unificazione politica e prima ancora fiscale, per non creare un'Europa a due o forse a tre velocità? la consapevolezza che un'armonizzazione, una semplificazione della fiscalità a livello sovranazionale, un contrasto deciso a livello europeo alle dinamiche della criminalità organizzata, che ribadisco essere la prima fonte di evasione,

una discussione che avrebbe contribuito a preparare una culla ben più confortevole per quell'Unione europea che di lì a poco sarebbe nata e che forse avrebbe meglio compensato quei sacrifici che il nostro e tanti altri Paesi europei hanno affrontato per realizzare quel progetto di cui solo adesso sembra si intuiscano le criticità. Non so dire se siamo ancora in tempo per recuperare questo ritardo, ma dato che ho sempre considerato l'esempio come prima fonte di stimolo per il cambiamento, rinnovo a lei, signor Presidente del Consiglio, l'invito che le feci un mese fa: l'Italia sia di esempio. Affrontiamo con convinzione le questioni che minano la credibilità del nostro Paese - corruzione, riciclaggio, evasione ed elusione fiscale anche in campo internazionale, reati contabili e la nostra azione persuasiva a livello europeo sarà incisiva e convincente, anche nei confronti degli Stati più dubbiosi. Abbiamo discusso, in questo periodo, decreti in cui sono state trattate emergenze di ogni tipo, vere o indotte: forse è il caso di dedicarci anche a quelle che abbiamo trascurato negli ultimi venti anni.

l'emergenza della disoccupazione giovanile in Europa. Condivido molto quello che ci ha detto, signor Presidente. Siamo consapevoli che nel nostro Paese la disoccupazione presenta diversi punti di emergenza: gli adulti che hanno perso il lavoro, i licenziati o le donne, giovani e meno giovani. Però, penso che sia arrivato il tempo di occuparsi, con misure specifiche, di giovani e di disoccupazione giovanile. C'è bisogno che ce ne facciamo carico; c'è bisogno di interventi specifici, perché rischiamo che, nella crisi più profonda del dopoguerra, alcune generazioni del nostro Paese non abbiano nessun contatto Il 22 aprile 2013 il Consiglio europeo ha emanato una serie di raccomandazioni relative all'istituzione della *Youth* *Guarantee*, in cui si riconosce che la disoccupazione giovanile lascia tracce permanenti, con rischi più pesanti di disoccupazione futura, con rischi di livelli di reddito ridotti in futuro e di trasmissione di povertà fra generazioni e con il consolidamento delle tendenze demografiche negative. negative. L'Europa propone uno strumento per contrastare questo quadro. Si dice che, entro quattro mesi dalla perdita di lavoro per un giovane fino a 25 anni

Per questo si stanziano 6 miliardi nel periodo 2014-2020. Noi, presidente Letta, sosteniamo e comprendiamo la sua richiesta di concentrare il più possibile le risorse e di poter cominciare ad utilizzarle già dall'inizio del 2014 e comprendiamo e condividiamo la richiesta di rifinanziamento a partire dal 2016. Bisognerà poi tener conto dei diversi sistemi nazionali e locali, delle differenze di genere o comunque delle differenze e della diversità dei giovani ai quali sono destinate le misure. Dobbiamo fare però delle cose fondamentali e generali per il nostro Paese. Bisogna riorganizzare i servizi per l'impiego; si tratta di riattivare la delega relativa ed esercitarla il prima possibile. Nel frattempo, però, bisogna collegare i servizi per l'impiego che ci sono, metterli in rete con i soggetti istituzionali e sociali coinvolti, anche per corrispondere alle richieste europee di presa in carico dei giovani. Poi bisognerà sviluppare la capacità di utilizzo dei diversi fondi europei in modo integrato. Non parlo solo del Fondo sociale europeo (c'è la proposta che, nell'ambito degli interventi finanziabili con il Fondo sociale, venga definita una specifica iniziativa a favore dell'occupazione giovanile), Parlo, ad esempio, del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (è essenziale il legame fra FSE e FESR per le nostre Regioni), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Insomma, bisogna lavorare in modo integrato. Poi, presidente Letta, noi abbiamo drammatiche disuguaglianze da colmare. Abbiamo le disuguaglianze territoriali (e qui bisogna essere consapevoli che, se cresce il Sud del Paese, le altre aree crescono di più), le disuguaglianze di genere (e qui fatemi dire che sta aumentando la povertà femminile ed infantile). Sappiamo tutti - e l'esperienza degli altri Paesi ce lo conferma - che le donne che lavorano fanno più figli e li allevano meglio. Abbiamo poi le disuguaglianze di reddito: rischiamo generazioni di uomini e donne da assistere, se continuiamo così. La lotta alle disuguaglianze genera coesione sociale e sviluppo, se la si affronta con spirito solidale. Nella *Youth* *Guarantee* si parla di esperienze di lavoro per i giovani. Da questo punto di vista, la situazione è molto pesante nel nostro Paese. Dovremmo trovare nuove possibilità, con progetti di interventi in ambiti caratterizzati da alta intensità di lavoro penso all'assistenza alle persone, all'intervento di ripristino ambientale e di cura del territorio, alla cura del patrimonio culturale e a molte altre cose che ci possono venire in mente - che permettano esperienze e messa alla prova delle competenze. Gli strumenti li abbiamo. Pensiamo all'esperienza del servizio civile: andrebbe adattata e rimodulata, ma ha già dato buona prova di sé. Bisogna tenere sempre presente, però, che non vanno mai svalutati il lavoro, le regole sottese al lavoro, la dignità dei giovani lavoratori. In effetti, si parla sempre di offerta qualitativamente valida. Ci sono poi la formazione e la lotta alla dispersione scolastica. Sono contenta della presenza della Ministra Bisognerà tener conto anche in questo caso delle differenze. I dati sulla dispersione scolastica ci dicono, ad esempio, che molti sono giovani stranieri; e sotto questo profilo va dato valore alla formazione, anche a quella professionale e tecnica. Occorrerà riqualificare scuole ed insegnanti. I nostri istituti tecnici hanno una grande tradizione

oltre a partecipare all'alleanza europea per l'apprendistato e a intervenire con modifiche alla normativa che rendano l'istituto appetibile in questo periodo di crisi, con l'apparato produttivo nella situazione che conosciamo, bisognerà integrare le diverse esperienze che sono già state sviluppate in diverse Regioni - presidente Letta, non credo di dover parlare a lei circa l'esperienza «Giovani Sìۚ» della Toscana - in cui, oltre a *stage* e tirocini, vengono incentivati progetti di lavoro autonomo e di autoimprenditorialità si dà supporto anche alla volontà di vita autonoma delle ragazze e dei ragazzi. Vanno valutate le esperienze fatte per coglierne gli aspetti positivi e i problemi che sono stati generati per superarli. Consiglio, siamo consapevoli che c'è bisogno di crescere e di riattivare la domanda interna per risolvere i problemi della disoccupazione. possa assolvere ad un compito fondamentale: non far sentire soli i giovani in una situazione così difficile, non abbandonarli e prepararli a cogliere con profitto i segnali, anche deboli, di una crescita che riparte. La sosteniamo, signor Presidente, perché crediamo che il Paese abbia bisogno della forza e dell'energia dei giovani e riteniamo che i giovani che vivono in Italia pensano, si sentono e si relazionano fra loro come giovani europei.

il Parlamento europeo riconosce la priorità della crisi climatica e della lotta al *global warming* per la salvaguardia del pianeta, per perseguire uno sviluppo sostenibile in termini di *carrying capacity*. Primario è dunque mantenere il riscaldamento del pianeta al di sotto dei due gradi centigradi. Ciò costituisce un'opportunità di cambiamento per definire nuove economie a basse emissioni di carbonio ed indurre una nuova rivoluzione industriale. Questo vincolo, signor Presidente, seppur imposto dalla preoccupazione per la salvaguardia del pianeta, rappresenta il motore di una nuova economia, in grado di dare risposte all'attuale crisi economica nel settore dell'energia, ma anche del turismo ecosostenibile. Nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza e del risparmio energetico, si giocherà, a livello planetario, la sfida dell'innovazione, della competitività, del lavoro e della capacità di futuro. Il modo in cui l'energia viene oggi impiegata non risponde a criteri di equità e sostenibilità: molti popoli non sono infatti ancora in grado di soddisfare i bisogni primari e le risorse appaiono già prossime al limite di sfruttamento. I dati provenienti da diverse fonti disponibili, istituzionali e non, sui *trend* occupazionali a livello internazionale, comunitario e nazionale, e le proiezioni al 2020, sebbene assai diversificati e non sempre confrontabili tra loro a causa delle diverse metodologie adottate, confermano una tendenza in atto incontrovertibile: la crescita di occupazione nei settori di nuova economia in grado di produrre un effetto compensativo rispetto a lavori tradizionali a forte impatto ambientale, ma di aprire prospettive occupazionali incoraggianti per fronteggiare l'attuale crisi e rilanciare l'economia mondiale. Da uno studio condotto dall'università Bocconi, congiunto al gestore dei servizi elettrici, si è visto che con lo sviluppo di tecnologie rinnovabili si porterebbe a 150.000 il numero degli occupati e soprattutto che, dallo sfruttamento del potenziale tecnologico, si prospetta la crescita occupazionale al 2020 di 250.000 È necessario investire in tecnologie che consentano un utilizzo razionale delle risorse disponibili a beneficio del maggior numero possibile di individui, nel rispetto dei limiti biofisici del pianeta. Crediamo sia necessario dare vita ad un nuovo patto per lo sviluppo, che assuma fra i suoi obiettivi prioritari un piano per la piena e buona occupazione giovanile e femminile in tutti i settori che abbiamo individuato far parte della *green economy*: diffusione dell'ecoinnovazione, risparmio energetico, sviluppo delle rinnovabili, riciclo della materia, tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, riqualificazione delle città, mobilità sostenibile. Innovazione, cultura ed economia sono soltanto degli *slogan*, ma rappresentano quella strategia concreta per un nuovo modello di sviluppo che il corso degli eventi ci suggerisce con buonsenso di intraprendere. Il Governo, le Regioni e gli enti locali devono coordinare le azioni, indirizzare le scelte e promuovere l'utilizzo di tali sistemi a favore dei cittadini. Utilizzare le fonti rinnovabili e ridurre i consumi energetici delle nostre abitazioni significa anche diminuire il costo delle bollette cittadini, sostenere tutte le famiglie in difficoltà, accrescere il *comfort* e valorizzare gli immobili, migliorare la qualità della nostra vita e del nostro ambiente con la riduzione dei consumi di combustibili fossili; in ultimo, ciò significa anche ridurre la dipendenza energetica dell'Italia. si dovrà passare necessariamente dalla diversificazione delle fonti energetiche e dall'uso delle rinnovabili, come è negli intenti delle direttive europee in tema di energia. Per questo, l'evoluzione del sistema elettrico nazionale passa obbligatoriamente dalla corretta pianificazione degli interventi di sviluppo della rete di distribuzione. Vorrei fare solo un accenno agli interventi ritenuti prioritari per il nostro territorio, in particolare a quelli finalizzati a permettere lo sviluppo delle reti nelle regioni insulari e isolate: mi riferisco al collegamento della Sicilia con la Calabria e al potenziamento delle reti a 380 e 220 con la realizzazione di un elettrodotto in doppio cavo sottomarino, ritenuto necessario non solo per garantire maggiore sicurezza del collegamento elettrico tra l'isola e l'area continentale, ma anche per incrementare gli scambi di energia tra le due zone, con evidenti benefici anche in termini di maggior concorrenza sul mercato energetico. Oggi siamo chiamati al rispetto dell'ambiente: teniamo in considerazione i cambiamenti climatici degli ultimi tempi, che hanno avuto effetti attesi anche nell'ambito del turismo. L'occupazione dei giovani può far ripartire tutto l'assetto occupazionale e va favorita con misure di accesso agevolato al credito e facilitazioni fiscali in grado di ridurre il costo del lavoro, senza però abbattere le retribuzioni. Occorre favorire la creazione di nuove imprese *green*, incentivando anche lo sviluppo del turismo ecosostenibile.

Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio dei ministri, onorevoli senatori, dopo un doveroso e deferente ricordo alla memoria del senatore Emilio Colombo, passo al confronto sulle comunicazioni che il Presidente del Consiglio ci ha reso sul prossimo Consiglio europeo, nel pieno rispetto del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 234 del 2012. Si tratta di una delle prime applicazioni di tale disciplina veramente innovativa rispetto al ruolo dei Parlamenti nazionali nella definizione della posizione nazionale in ambito europeo; norma per cui mi ero battuto con successo nella scorsa legislatura in ricezione delle indicazioni che nascevano dal Trattato di Lisbona. Tale procedura valorizza in modo significativo il confronto Parlamento-Governo e a mio parere potrà rappresentare il riflesso politico-istituzionale del concreto atteggiarsi delle forze politiche che sostengono il Governo. In particolare, apprezzo l'obiettivo di ricercare una posizione condivisa su rilevanti questioni come il sostegno alla crescita economica, la lotta alla disoccupazione giovanile, l'unione bancaria e la tutela del risparmiatore. Il mio plauso si indirizza soprattutto al Presidente del Consiglio che, con il suo intervento, segna al contempo un'apprezzabile continuità e un'altrettanto apprezzabile discontinuità. Sotto il primo profilo, si prosegue, come già per l'intervento del 22 maggio scorso, nel solco delle iniziative del Governo Monti e del ministro Moavero, nel raccordare con procedure parlamentari «forti» e impegnative il lavoro e l'impegno dell'Esecutivo nelle sedi comunitarie. La discontinuità, invece, si avverte rispetto ad una consuetudine che vedeva in anni passati la materia europea relegata ad un ruolo secondario, frutto di decisioni e indirizzi nati fuori dal contesto politico nazionale, salvo poi invocare la natura «matrigna» dell'Unione, a causa di orientamenti sostanzialmente Riprendendo la felice distinzione dello stesso presidente Letta nel suo discorso di insediamento, questo è un chiaro indirizzo di politica. Quanto invece alle politiche, rimarco, da presidente della Commissione finanze e tesoro, la qualità e la rilevanza delle questioni oggetto del prossimo Consiglio. Mi preme, peraltro, premettere ancora una considerazione di fondo: al di là delle singole materie all'ordine del giorno della riunione di Capi di Stato e di Governo, appare di tutta evidenza che l'obiettivo degli incontri futuri non può che essere la definizione di strategie complessive e di strumenti adeguati per affrontare la grave recessione in atto e riportare i livelli produttivi dell'area comunitaria su *standard* precrisi. Le prospettive finanziarie presentano oggi un grado minore di incertezza rispetto al passato e quindi le scelte della politica possono orientare complessivamente l'azione dei Governi in una direzione che può giovarsi delle conquiste sul fronte del rigore finanziario, che rimane un orizzonte imprescindibile, ma non più come l'unica strada da percorrere. La politica fiscale e tributaria è il centro dell'attuale decisione politica: va rimarcato il ruolo propulsivo delle politiche fiscali. Occorre individuare i settori per i quali il livello del prelievo ostacola la crescita economica e operare di conseguenza. Non si tratta di scegliere i comparti produttivi meritevoli di attenzione, ma di indirizzare le risorse pubbliche a favore delle attività orientate al mercato, penalizzando - anche attraverso un incremento delle tasse - le posizioni di rendita e di ricchezza improduttiva. A me pare che l'attuale crisi si manifesti non solo con la contrapposizione tra protetti e non protetti, tra vecchi e giovani, tra donne e precari e integrati, ma sopratutto tra chi opera nel contesto della concorrenza e nel mercato (anche globale), e che quindi è costretto a recuperare competitività ed efficienza, e chi non è esposto a tale rischio. Il fisco, quindi, deve orientarsi verso il primo settore, anche con un'azione di semplificazione e snellimento delle procedure. Auspico pertanto che tale impostazione, nel rispetto dei patti sottoscritti, ma nella convinzione di operare per una più elastica applicazione dei vincoli comunitari, sia alla base della discussione del Governo italiano per il prossimo Consiglio. Oltre a tale impostazione di fondo, voglio svolgere alcune considerazioni di merito rispetto alle questioni oggetto del Consiglio europeo. Per quanto riguarda le raccomandazioni all'Italia, la Commissione si sofferma, tra l'altro, sulla dichiarazione resa dal Governo italiano il 17 maggio, volta a confermare gli impegni assunti con il Programma di stabilità 2013 e ad annunciare nuove misure da adottare nel pieno rispetto degli obiettivi di bilancio. Tali misure, contenute nel decreto legge n. 54 del 2013, comprendono la sospensione della rata di giugno dell'IMU sulle abitazioni occupate dal loro proprietario proprietario (cosiddetta IMU prima casa), e il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali attraverso una riallocazione delle risorse di bilancio disponibili oltre a quelle congelate in occasione della riforma del mercato del lavoro nel 2012. Secondo la valutazione della Commissione, tali misure, se attuate in modo coerente, «non hanno un'incidenza significativa sul *deficit»*, che dovrebbe rimanere inferiore al valore di riferimento del 3 per La Camera ha già licenziato il testo del decreto-legge e le Commissioni riunite 6a e 11a del Senato si apprestano ad esaminare tale provvedimento: senza anticipare l'esito del dibattito - che è rimesso alle rispettive Commissioni - esprimo l'impegno a convertire il decreto in tempi rapidi per confermare gli impegni assunti dall'Italia su tale fronte. Il rinvio del pagamento della rata dell'IMU non è un *escamotage*, ma serve al Governo e al Parlamento per individuare la soluzione condivisa più adatta su un fronte fiscale che vede allineate diverse opzioni: nel corso delle audizioni dell'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili, il cui ciclo si è concluso oggi in Commissione finanze e tesoro, sono emersi molteplici spunti e differenti posizioni, ma appare confermata la strada di una revisione della disciplina fiscale in grado di ridurre considerevolmente il prelievo. Anticipo peraltro che una revisione dell'IMU va inquadrata in un disegno complessivo di riforma della tassazione sugli immobili: in tale quadro andranno quindi valutate le scelte - anche in vista di interventi di compensazione e per equilibri differenti - che si andranno a compiere sul comparto.

primo obiettivo è la firma di un patto precostituzionale da parte dei Paesi dell'eurozona, che contenga l'impegno di passare da un Governo provvisorio ed intergovernativo ad uno democratico e federale, della moneta, della fiscalità dell'eurozona e dell'economia; obiettivo è la convocazione in tempi brevi di una Convenzione costituente europea con il mandato di elaborare la Costituzione federale dell'Unione e di stabilire le norme transitorie per regolare le relazioni e il passaggio fra vecchie e nuove istituzioni europee. Solo così avremo contro l'Europa delle tecnocrazie, la vera Europa dei popoli e avremo argomenti per vincere troppo facili demagogie. Buon lavoro, signor Presidente.

istituzionale che intellettuale. La sua lezione non è solo politica e rimane a tutti. Egregio Presidente del Consiglio, abbiamo apprezzato particolarmente il suo intervento per l'estrema concretezza che lo contraddistingue, come sempre peraltro. Lei ha fatto riferimento alla risoluzione del 21 maggio e puntualmente è venuto qui, in quest'Aula, a rendere conto di ciò che è stato fatto e a confermare anche la linea politica che il Parlamento le le ha indicato e che lei con il suo Governo sta seguendo. Abbiamo apprezzato anche le due emergenze da lei delineate: quella dell'occupazione giovanile e quella della politica economica. Lei stesso ha citato dati

ne va di mezzo il capitale umano rappresentato dai giovani e quindi ne va di mezzo la futura classe dirigente. Ci giochiamo tutto su questa sfida. Quindi, apprezziamo particolarmente il fatto che lei l'abbia considerata come la sfida cruciale

dare garanzie anche con regole nuove. Lei ha giustamente parlato di un mercato del lavoro più flessibile e più mobile; ha parlato addirittura di un mercato unico del lavoro: questo è un obiettivo sicuramente difficile, ma ineludibile.

ad essere competitivi. Dobbiamo creare anche altre condizioni, ad esempio aumentare la conoscenza delle lingue. È impensabile che un giovane, ma non solo, possa cambiare lavoro o muoversi per il mondo se non conosce le lingue. E l'Italia è drammaticamente indietro da questo In altri Paesi europei i giovani conoscono due o tre lingue, a volte anche quattro, si muovono agevolmente dalla sera alla mattina e se perdono il lavoro si spostano e ne trovano un altro.

Purtroppo, la scuola è bloccata, dobbiamo dirlo. Il mondo cambia a ritmi vertiginosi e la scuola dovrebbe cambiare e adeguarsi velocemente. Invece, oggi abbiamo una scuola bloccata e ogni volta che si tocca qualcosa succede il finimondo. che dovremmo imparare a concepire l'istituzione scolastica non solo come un insieme di insegnanti, di diritti e di contratti, ma come una istituzione che prepara il cittadino, che lo segue, una istituzione che accompagna l'evoluzione dei tempi.

portato ad ottimi risultati che, purtroppo, in Italia ancora non abbiamo. Abbiamo condiviso anche le sue parole forti in merito ad una scelta identitaria, una scelta dirimente, che è quella che farà la differenza. Siamo molto contenti

Così come condividiamo la sua convinzione di pensare a risultati concreti, di darsi delle scadenze. Lei ha parlato del 1° gennaio 2014, di stanziamenti calibrati con gli anni e con i tempi. Sono sicuro che lei

(come lei stesso ha detto bene), investimenti sul credito. Non si può creare un'azienda, non si può investire se non si hanno le risorse. I giovani oggi non sono in grado di fornire alle banche le garanzie per ottenere le risorse necessarie. Quindi, questo sforzo particolare sul credito, sulle banche attente al territorio, su quelle che investono sul territorio oggi è assolutamente indispensabile. Anche il ruolo maggiormente incisivo

Concludo ringraziandola per la sua convinzione che ha espresso anche in quest'Aula, per aver parlato di scelte non al ribasso ma viceversa di una sfida, di un rilancio forte; per aver dimostrato di credere, per aver parlato dell'Europa dei popoli, dei cittadini e delle menti. Spero davvero che questa sua questa sua ambizione, che esprime anche a nome del Parlamento intero (ma vorrei dire di tutto il popolo italiano, il quale ha sempre creduto nell'Unione europea, e il nostro Paese è stato tra i fondatori

ricordava quelli che definì i tanti Soloni europei e la centralità della formazione degli Stati Uniti d'Europa esattamente come il primo fra tutti gli obiettivi politici da raggiungere. Vogliamo salutare e ricordare il senatore e naturalmente ringraziarlo per aver speso una vita intera per la Repubblica italiana. Signor Presidente del Consiglio, sappiamo che le prossime riunioni del Consiglio europeo porranno - come lei ha ricordato stasera - al centro dell'agenda, oltre ai consueti obiettivi della competitività, della crescita e del percorso di completamento dell'unione fiscale e monetaria, la valutazione di uno sforzo per affrontare la questione della disoccupazione giovanile. È un tema che un tema che naturalmente anche a noi sembra di grande interesse, anche perché (è stato detto), per le dimensioni che ha assunto, è urgente ormai anche solo nominare la questione della disoccupazione che colpisce le giovani generazioni, in particolar modo da quando si è aggravata la crisi, anche - occorre dirlo - per le misure procicliche suggerite dalle istituzioni europee e adottate dai Paesi della zona euro. Per questo, signor Presidente, condividiamo lo sforzo che lei sta sostenendo nel far diventare queste questioni almeno un terreno di discussione collettiva. A noi però che le misure in esame richiedano una qualche ulteriore a partire dalle osservazioni circa i provvedimenti da adottare per rafforzare la competitività e la crescita. Ebbene, nei cinque anni che abbiamo alle spalle e che hanno visto prima esordire e poi approfondirsi la crisi gravissima delle economie mondiali e in special modo europea, i termini «competitività» e «crescita» sono stati un mantra che abbiamo ascoltato regolarmente ad ogni vertice. Ma le misure che sono state suggerite e adottate ci sembrano non aver stimolato né la competitività ma né la crescita. Anzi, si sono indebolite le economie, colpite da quelle misure che, con un vero e proprio ossimoro, sono state definite di «austerità espansiva». Come però è reso evidente da tutti gli indicatori, di espansivo c'è ben poco. Non solo non si è posto rimedio al problema del debito pubblico, ma - come anche nel caso italiano - per effetto dell'austerità peggiorano gli indicatori economici ed è in particolar modo colpita l'occupazione, innanzitutto quella giovanile. E non voglio ripetere in questa sede i dati ISTAT, che lei ha già ricordato, le drammatiche cifre che parlano ormai di una questione inedita e, per l'appunto, drammatica. Noi pensiamo, insieme alla CGIL, che le politiche attive del lavoro debbano rimanere competenza del settore pubblico; ma il settore pubblico, però, è quello più falcidiato dalle politiche di riforma strutturale che ancora si ritiene da troppi debbano essere l'alfa e l'omega

che ha favorito l'ulteriore frammentazione e precarizzazione del lavoro senza offrire nessuna contropartita seria e tantomeno rafforzare il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Intendiamoci, noi apprezziamo e vediamo con favore gli strumenti volti a favorire 1'occupazione giovanile come la *Youth Guarantee*. Strumenti come questi costituiscono un primo passo per affrontare la questione della disoccupazione giovanile che emerge ormai purtroppo come un problema strutturale. Ma lo riteniamo però un primo passo insufficiente, soprattutto per l'esiguità delle risorse stanziate. Ci sembra evidente che è proprio il taglio delle risorse pubbliche che le rigide regole dell'austerità impongono a mettere a rischio l'efficacia di questi programmi. Per questo ci sembra insufficiente che tra le priorità si ponga la questione dell'unione fiscale e bancaria, che rischia di rimanere monca perché priva di una corrispettiva unione economica e politica. Rispetto ai pur apprezzabili e condivisibili propositi di rafforzare la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, traslare sempre più la tassazione dai fattori produttivi ai patrimoni e ai consumi, nonché la raccomandazione a a procedere alle semplificazioni dell'apparato amministrativo, si riscontrano però non pochi limiti, e poche e insufficienti sembrano le misure in grado di invertire la rotta. Nessun riferimento viene fatto, invece, alla priorità della lotta ai paradisi fiscali, verso cui, come sappiamo, si dirotta una buona quota dei grandi redditi generati in Europa, e a forme di disincentivazione attraverso la tassazione coordinata delle traslazioni bancarie. Oppure, in tema di occupazione, è un bene che si faccia riferimento alla decontribuzione per i neoassunti, ma andrebbe finalizzata alla stabilizzazione del rapporto di lavoro e non solo ai fini della riduzione della imposizione fiscale per le aziende. In definitiva, vorremmo dirla così. A noi sembra che il complesso dell'agenda del prossimo Consiglio europeo sia ancora troppo interna al perimetro dell'austerità che ha segnato la politica delle istituzioni europee nel corso di tutta la gestione della crisi e che l'esiguità delle risorse stanziate e rese disponibili, il *credit crunch* che ancora soffoca soprattutto le piccole e medie imprese e le politiche procicliche messe in atto dai Governi, mettano seriamente a rischio il raggiungimento di quei pur minimi obiettivi che il Consiglio si è dato. Proprio per questo anche noi pensiamo che le raccomandazioni rivolte dal Consiglio europeo dopo l'uscita del nostro Paese dalla procedura di infrazione non ci consentano sufficientemente di riattivare la nostra economia. E non sembrano neanche tenere conto di quelle dichiarazioni provenienti dallo stesso Fondo monetario internazionale che mettono sotto accusa finalmente le politiche recessive, ritenendole per la prima volta, senza mezzi termini, inadeguate a portare l'economia europea fuori dalla crisi, e anzi causa della spirale recessiva che che attanaglia l'Europa. Per questo è evidente che anche il problema della disoccupazione, e della disoccupazione giovanile in particolare, non può essere slegato dalla questione delle regole di bilancio e della politica di austerità:

con uno zelo davvero eccessivo, il *fiscal compact* e l'obbligo di pareggio di bilancio in Costituzione, non essendo tra l'altro gli Stati affatto obbligati, ma solo facoltizzati a rendere norma costituzionale quello che è un Trattato tra Stati. In tal modo si è costituzionalizzata l'austerità, che è una politica economica e per di più, secondo noi, una politica sbagliata. Né tantomeno il DEF 2013 sembra lasciare spazio a spiragli che consentano di uscire dalla rigida gabbia della sostenibilità finanziaria, ma rimane ancorato alla prospettiva del pareggio strutturale di bilancio per il 2014-2015 e su previsioni di crescita del PIL irrealistiche, che non consentono nessuna possibilità di mettere in campo una politica economica anticiclica.

prioritariamente quello definito dal Patto di stabilità e crescita, laddove si guarda purtroppo solo alla stabilità e poco alla crescita, sia un grave errore; e che, se la miopia delle *leadership* europee si prolungasse ancora, provocherebbe conseguenze disastrose, che renderebbero vani tutti gli sforzi per invertire o rendere anche solo meno duri gli effetti della più lunga crisi che l'Europa abbia mai conosciuto. Signora Presidente, colleghe e colleghi, signor Presidente del Consiglio, lei oggi ha già ascoltato molti consigli e molte precisazioni, quindi la la vorrei distrarre con un solo numero, diffuso oggi, che trovo significativo, e con un breve ragionamento che vorrei condividere con lei, più sull'approccio che non sulle tematiche specifiche. Il numero che oggi mi ha colpito è per cento di consumi alimentari in aprile. Domani in quest'Aula discuteremo anche su mozioni che riguardano la povertà, e credo che questo numero diventi significativo anche per lei, per i termini di confronto che dovrà avere con i nostri *partner* europei, perché questa poi è la realtà. Lei inoltre ha citato, come molti colleghi, anche i numeri specifici. La disoccupazione la conosciamo tutti, purtroppo.

onorevole Letta, non è l'Europa che si immaginavano Schuman, De Gasperi, Adenauer e, probabilmente, non è nemmeno la stessa Europa che si immaginava il presidente Colombo, che oggi

perché hanno una cultura politica diversa. Allora, presidente Letta, se c'è una cultura politica da mettere a disposizione, mettiamola a disposizione e confrontiamoci con quelle culture politiche che, ancora diverse dalla nostra, non hanno forse la stessa interpretazione di Europa. Europa. Finché non raggiungeremo quella sintesi vera con le altre culture politiche europee, infatti, difficilmente riusciremo ad immaginarci un'Europa che abbia quell'anima che stiamo ricercando. Quando parlo di mancanza d'anima, mi riferisco anche a quel dissolvimento, almeno apparente, delle nostre storie, della storia dei nostri territori, della storia di quelle sensibilità sociali che non sono più così riconosciute e riconoscibili. Si tratta di quella forma di mancanza di impegno politico che, a volte, guardando i semplici numeri dell'Europa, ci fa immaginare che in quei numeri ci siano per forza delle realtà. realtà. Le dico un'altra cosa, signor Presidente: ci è uno Stato, all'interno di questa Europa, che un po' troppo spesso fa il padrone di casa. Richiamo un dato che viene dagli atti parlamentari, e che ricordano anche i colleghi che frequentavano le Commissioni affari costituzionali e bilancio quando si parlò del pareggio di bilancio. Ebbene, un passaggio è evidente.

Paese pensi di scaricare delle responsabilità sugli altri Paesi; e non ci piace immaginare che in quei Paesi si possa salvare quello che si ha in casa (e mi riferisco proprio alla Germania) creando dei conflitti sociali. I conflitti sociali non possono più essere di moda. Non lo sono più.

assolutamente interclassista. Questo è un vecchio termine, che però è utilizzato oggi da qualcuno per spiegare che nessuno si salva: non si salva l'artigiano, purtroppo, non si salva l'operaio e non si salva l'industriale. *(Applausi della crisi ha una sola risposta: ritrovare quella forma di collaborazione che consente, con la stessa forma d'interclassismo, di rispondere in maniera concreta a questo tipo di crisi. Questo dobbiamo rappresentare all'Europa. Noi la vogliamo poi sollecitare su un'altra questione, che riteniamo sia quella concreta. È non è l'immagine del Nord contro il Sud e dell'egoismo, ma è l'immagine di una realtà politica e di una realtà economica e sociale. una guerra fra Nord e Sud, ma queste sono realtà diverse. Purtroppo al Nord, e lei lo sa, il motore si sta spegnendo e nel momento in cui si dovesse spegnere il problema ci riguarderà tutti. Ma vogliamo essere propositivi, signor Presidente. Quando noi le proponiamo un'idea di macroregionalità in Europa e anche nello Stato stesso, le vogliamo rappresentare qualcosa che riguarda l'omogeneità sociale ed economica dei territori. Lei che ha una storia politica sa benissimo che a livello nazionale non è più applicabile un'unica politica di coesione economica e sociale. Possono rimanere i principi ma non può esserci un'unica soluzione, perché i territori hanno vocazioni diverse, hanno storie diverse, hanno problemi diversi. riusciamo, anche attraverso la collaborazione con questo Governo, a far capire che l'Europa ha la possibilità di aiutare delle situazioni omogenee, dove si rimettono allo stesso tavolo tutti gli attori sociali insieme al credito, insieme agli enti locali, insieme alle organizzazioni sindacali, su quei territori, con quelle particolarità, si può creare qualcosa di nuovo per rilanciare, a livello nazionale, un'idea di economia sostenibile e diversificata a seconda delle valorizzazioni che si possono dare ai territori e, a livello europeo, la credibilità e la riconoscibilità di quei territori con una nuova Europa. Allora, forse riusciamo a dare un nuovo indirizzo. Questa è la nostra idea originale.

Quella rappresentazione che lei dovrà fare del nostro Paese in un contesto difficile può avere il sostegno di tutti, però deve esserci anche quello spazio politico che consenta a noi tutti di riconoscerci in quell'azione verso

fosse un semestre che porti sentimenti e idee, e non solo numeri. *(Applausi Presidente, onorevoli colleghi, io e tutti i componenti del Movimento 5 Stelle ci uniamo al cordoglio per la scomparsa del senatore Emilio Colombo e ci tengo a ribadire, personalmente, la grande emozione che provai il primo giorno entrando in quest'Aula nel vedere lì davanti l'ultimo Padre costituente. Presidente, in una situazione di emergenza come l'attuale, sarebbe auspicabile realizzare una riforma finanziaria che sia etica e che produca a sua volta una riforma economica e salutare per tutti. Oggi c'è uno squilibrio negli investimenti finanziari per cui, a fronte di grandi riunioni internazionali, si muore di fame. Nell'attuale crisi economica il reddito di una minoranza cresce in maniera esponenziale, mentre quello della maggioranza si indebolisce. Questo squilibrio deriva da ideologie che promuovono l'autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria, negando così il diritto di controllo degli Stati, pur incaricati di provvedere al bene comune. Queste parole sono state pronunciate da una persona nuova e rivoluzionaria e, badate bene, non è quel provocatore di Beppe Grillo, ma è Papa Francesco. La povertà è la condizione di singole persone o collettività umane che si ritrovano ad avere, per ragioni di ordine economico, un limitato o del tutto mancante accesso a beni essenziali. Povertà è anche quella cosa che ti fa scegliere se morire di stenti e umiliazione per mancanza di lavoro o decidere di lavorare in un luogo malsano, per morire poi di cancro, come a Porto Marghera o all'ILVA di Taranto. Ma la povertà è anche la fame di essere amati (come diceva madre Teresa di Calcutta ), il bisogno di essere accolti, protetti, difesi, considerati. In Italia la povertà sta crescendo, e non solo quella economica. Redditi e condizioni di vita, persone senza fissa dimora, consumi sempre più contratti, assenza di lavoro registrano numeri sempre più allarmanti; un dato per tutti: in Italia solamente i bambini poveri sono quasi 2 milioni. Definiamo come poveri coloro che non possono sostenere spese inaspettate, che non possono onorare il mutuo della casa, che non riescono a far studiare i propri figli, che non possono permettersi pasti adeguati ogni due giorni, che non riescono a pagare più le bollette di luce e gas. Anche se sembra assurdo ricordarlo, una delle gioie più grandi per una persona con problemi economici è avere una casa riscaldata nel freddo inverno e potersi lavare con l'acqua calda. È una sensazione di conquista che chi non l'ha provata non può comprendere e parlarne qua, tra velluti damascati, auto blu, privilegi di casta e lustrini, lo so, può sembrare una missione quasi impossibile, e non vorrei che questi momenti andassero perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. George Farquhar scriveva: «Nessun crimine è vergognoso quanto la povertà». Ebbene, arrivano nuove forme di suicidio mai viste in Italia. Presidente Letta, oggi le persone arrivano a darsi fuoco. Decidere di immolarsi col fuoco è l'atto estremo; darsi fuoco è una denuncia, una denuncia politica. Sembrano bollettini di guerra: un uomo si impicca perché senza lavoro; un uomo non viene pagato da due anni e si dà fuoco; marito e moglie si suicidano per stenti e il fratello di lei si uccide; un imprenditore si spara alla testa e potremmo continuare all'infinito. Il *welfare* che poggia sulla famiglia, come ammortizzatore sociale è un fallimento: la famiglia oggi non ce la fa più. I vecchi con le loro sempre più misere pensioni devono mantenere i figli giovani e meno giovani, disoccupati e inoccupati, che nemmeno lo cercano più il lavoro perché, tanto si sa, il lavoro non c'è e se va bene diventi uno dei tanti nuovi schiavi cui viene rubato il tempo, magari in un *call center* a 500 euro al mese senza garanzie per il futuro. Fino a quando questo miserevole equilibrio potrà funzionare? Signori, siamo lo Stato, siamo noi che decidiamo per il bene o il male dei cittadini. Nessuno vuole la sofferenza e nessuno si deve sottrarre alle proprie responsabilità: sono le scelte che rivoluzionano le cose. Partiamo pure dal concetto che i soldi non spariscono, ma semplicemente si spostano e abbiamo il dovere di spostarli là dove sono le emergenze. Vogliamo avvicinarci all'Europa? Ebbene, noi del Movimento 5 Stelle chiediamo ad alta voce che venga istituito il reddito di cittadinanza, perché nessuno deve rimanere indietro perché siamo obbligati a fare un qualcosa che avvicini le persone allo Stato, uno Stato che dovrebbe far sentire le persone difese accudite e benvolute. Evitiamo le ulteriori umiliazioni delle carte di povertà (voi le chiamate *social card*)*.* Avete mai avuto l'ebbrezza di possedere una carta del genere? Avete mai provato l'umiliazione di chi va alla cassa di un supermercato e fa di tutto perché il vicino non veda come sta pagando la spesa? Reddito Reddito di cittadinanza, non significa attuare politiche assistenziali, ma significa dare corpo al principio di eguaglianza sostanziale, sancito nella nostra Costituzione all'articolo 3, dove i padri e madri costituenti avevano previsto che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Popolo della Libertà rivolgo un commosso omaggio alla memoria di Emilio Colombo. Per ragioni anagrafiche ho avuto l'occasione di conoscerlo e di frequentarlo tantissimi anni fa.

seguendo attentamente il dibattito, dando a tutti noi una lezione che credo dobbiamo ricordare. lei ci ha fatto un discorso serio e concreto. La situazione economica è drammatica: la gente e l'opinione pubblica reagiscono con rabbia quando discutiamo e facciamo polemiche su argomenti che non riguardano l'economia. È importantissimo che il Governo e il Parlamento dicano con chiarezza, attraverso parole semplici, che cosa si fa, come e in quali tempi. Non si possono fare tutte le leggi in pochi giorni, ma tracciare un percorso certo nei modi e nei tempi si può e si deve fare. La connessione tra l'economia e l'Europa è strettissima. Non c'è dubbio che un motivo non secondario secondario della nostra crisi risiede nel fatto che, fin dal 2008, molti Paesi extraeuropei si sono concentrati sullo sviluppo, mentre noi in Europa abbiamo pensato soprattutto al contenimento del *deficit* e solo di recente ci siamo concentrati sullo sviluppo. Lo sviluppo si realizza attraverso una serie di azioni diverse, che si ispirino tutte ad un' unica filosofia. Desidererei soffermarmi su due degli argomenti specifici oggetto della riunione europea dei prossimi giorni, il primo

La BCE non può stampare moneta: nel frattempo, Stati Uniti d'America e Giappone stampavano moneta. Il Fondo monetario internazionale di recente ha suscitato scalpore dicendo che forse aveva sbagliato atteggiamento con la Grecia, mentre i cittadini greci hanno sofferto e continuano soffrire pene sociali indicibili. Nel settembre del 2008 vi è stata la crisi della Lehman Brothers. Pochi giorni dopo, ai primi di ottobre, a Parigi si sono riuniti l'Italia, la Francia, la Germania e l'Inghilterra insieme ai vertici dell'Europa: desideravano trovare un accordo su come sostenere il sistema bancario europeo. La conclusione fu: ciascun Paese faccia quello che ritiene di fare. Non ci fu cioè nessun tipo di unione in questo settore. Nel giugno 2010 la crisi è passata dal sistema bancario al sistema dell'indebitamento pubblico: anche qui l'Europa ha lasciato ogni Paese a risolvere i propri problemi. Solo nel 2012 - e per fortuna nel 2011 a Trichet era subentrato Draghi - la BCE è intervenuta ad aiutare alcuni dei nostri Stati. Gli aiuti alle banche non sono andati a vantaggio dei loro clienti; anzi, i vari Basilea 1, 2 e 3, ponendo vincoli alle banche, in realtà hanno fatto si che le banche nei confronti dei loro clienti fossero più fiscali e meno disponibili ad elargire moneta. Questa è una motivazione grandissima della crisi alla quale noi stiamo assistendo, così come si è determinata. Bisogna adesso che si realizzi assolutamente una vera unione bancaria che garantisca solidità e trasparenza al sistema e che faccia sì che alle famiglie e alle imprese vengano concessi crediti. Passiamo ai giovani. Da quando vi è stata l'industrializzazione, cioè per più di un secolo, abbiamo visto che i figli guadagnavano più dei loro genitori spesso li aiutavano. Negli ultimi anni, prima i figli hanno cominciato a guadagnare meno dei loro genitori e, adesso, non trovano più posti di lavoro. Questa è la situazione nella quale ci troviamo. Signor Presidente, è molto opportuno che domani il Consiglio dei ministri adotti provvedimenti concreti a favore dei giovani; è opportuno per i nostri giovani e per il nostro Paese ed è opportuno perché lei sarà più forte nel fare delle richieste specifiche all'Europa sull'argomento. Ecco, io non penso di uscire dall'argomento se dico che i giovani meritano anche che, nei loro confronti e nei confronti della società, ci sia l'affermazione di valori morali e ci sia l'affermazione che gli squilibri sociali non debbono essere eccessivi. essere eccessivi. La settimana scorsa, il Senato ha approvato quasi all'unanimità (c'è stata l'astensione da parte di qualcuno) una mozione che detta le linee al Governo per le nomine che questo dovrà fare negli enti pubblici o nelle società in cui lo Stato abbia una partecipazione rilevante. Una di queste norme prevede una limitazione degli emolumenti. Abbiamo votato tale norma con qualche preoccupazione, perché se da una parte è giusto porre un limite, dall'altra c'è la preoccupazione che anche nelle aziende a partecipazione pubblica importanti vi siano *manager* di rilievo. Io ho un'età avanzata e ricordo che, quando ero giovane, un *manager*

L'obiettivo che si prefiggeva, uno dei vanti della FIAT, era che ogni anno si aumentasse l'occupazione. Ebbene, Vittorio Valletta era un *manager* che aveva un grande potere,

signor Presidente, che se l'Europa si ponesse l'obiettivo di prevedere una limitazione a livello europeo, per poi farsene interprete a livello di G20,

innescheranno un meccanismo virtuoso che produrrà risultati concreti, che sono indispensabili, ed invertirà una situazione psicologica drammatica nella quale ci troviamo, ridando finalmente a questo nostro Paese e alla nostra Europa la prospettiva che uno sviluppo è possibile.

inizio anch'io con un doveroso ricordo del presidente Colombo per la sua preziosa testimonianza di vita, ed entro subito nel merito. Presidente Letta, sono convinto, dopo l'intervento che lei ha fatto oggi in che l'Italia potrà presentarsi a testa alta al prossimo Consiglio europeo, non solo per le proposte che lei porterà, ma anche in virtù delle azioni di risanamento realizzate nei conti pubblici negli ultimi due anni

sui mercati a livello internazionale e darà all'Italia una maggiore capacità di incidere sulle politiche dell'Unione. Ricordiamo però che questo è un risultato frutto di un'austerità pesante, di un rigore sui conti pubblici che ha richiesto ingenti sacrifici alle famiglie, alle imprese, ai cittadini, in particolare quelli a più basso reddito. Oggi il Paese è in grande difficoltà, con aziende grandi e piccole che chiudono, una pressione fiscale troppo elevata, una disoccupazione allarmante. In queste settimane lei ha molto positivamente portato all'attenzione dei nostri *partner* europei la difficile situazione dell'occupazione, di quella giovanile in particolare, che è italiana ma comune anche a molti altri Paesi europei e richiede immediate misure da parte dell'Unione. È quindi importante spendere ora nel Consiglio europeo questa credibilità per impegnare la Commissione ad attuare interventi più decisi di dare nuovo ossigeno alle imprese, ai disoccupati e ai giovani italiani. Oggi dobbiamo mettere al centro il tema della crescita e dell'occupazione. Solo un'avvertenza: non facciamoci attrarre dall'accattivante suggestione di poter sforare il parametro del 3 per cento nel rapporto tra *deficit* e PIL. Forse è vero, come qualcuno ha detto, che anche facendolo non saremmo cacciati dall'Europa, di cui siamo orgogliosi fondatori, ma il tema è un altro e riguarda il modo in cui vogliamo stare in Europa: non come fanalino di coda, non come anello debole, nazione inaffidabile; vogliamo essere il motore del cambiamento della politica europea, e questo lo si ottiene solo partendo dal rispetto dei patti. dei patti. Oltre al tema dell'occupazione, su cui lei si è intrattenuto e rispetto al quale anche il dibattito è stato molto esplicito, chiediamo di cambiare passo per quanto riguarda la politica economica in senso più specifico. Noi individuiamo alcuni passaggi su cui vorrei soffermarmi. Innanzitutto, come diceva nel suo intervento, occorre un'attuazione più incisiva del programma europeo sulla crescita e l'occupazione, fondata su un ruolo più forte della Banca europea per gli investimenti, per favorire il credito che, come sappiamo, è motore dello sviluppo. secondo luogo, credo andrebbe riproposto in Europa il rilancio di un piano di grandi infrastrutture europee con l'emissione di *project bond* garantiti da obbligazioni di tipo europeo: questo è un tema abbandonato, ma credo che per lo sviluppo sarebbe importante riproporlo.

infrastrutture, ricerca, formazione, politiche di sviluppo settoriale oltre che dell'occupazione. Mi auguro che l'Italia abbia la forza di porre tale tema in questo Consiglio europeo, significherebbe poter disporre nel 2014 di margini di flessibilità importanti, che potrebbero permettere di riconsiderare il Patto di stabilità interno per i Comuni e anche la conclusione già nel 2014 del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese.

sugli obiettivi di crescita degli investimenti per il sistema dell'occupazione, della ricerca, della capacità di creare sviluppo. ad esempio, che ciò da noi significherebbe che il Fondo sociale potrebbe diventare nei sei anni che abbiamo di fronte il vero motore di una politica per l'occupazione e per i giovani. Concludendo, signor Presidente, le rivolgo un ultimo incoraggiamento a proseguire nella sua azione decisa in Europa. Le istituzioni europee non siano solo i luoghi della ragioneria e della finanza: gli accordi di stabilità sono strumenti, non il fine; il fine di un progetto europeo è fatto di lavoro, crescita, inclusione sociale. Prima delle tabelle e dei numeri dei vincoli macroeconomici che ci legano ai nostri *partner* ci sono i comuni valori che condividiamo, i quali ci portano a dire che vogliamo stare in Europa con una vocazione italiana a essere motori di un'integrazione europea più portatrice di opportunità positive e socialmente avanzate per tutti i suoi concittadini. In questo senso le auguro buon lavoro per il nostro Paese e per l'Europa unita.

questo tipo di dibattito è oggi un'innovazione molto importante, che è iniziata qualche mese fa, e che sicuramente darà, a chi giovedì dovrà andare a sedersi attorno a quel tavolo - nel quale bisogna rappresentare con una sola persona un intero Paese - una forza maggiore, una consapevolezza diversa rispetto alla capacità di far sì che sui temi principali dei quali si parlerà il Parlamento italiano, cioè il luogo della sovranità popolare,

fondamentale, e io vi ringrazio delle parole che sono state dette e che sicuramente mi rendono oggi maggiormente in grado di affrontare questo tema, tra l'altro,

non può che uscire dalle istituzioni europee; quindi, il Consiglio europeo è il luogo nel quale tutto ciò deve avvenire, sapendo che la crisi non è limitata ad uno o più Paesi: è una crisi di tutti,

Vedere ancora oggi la difficoltà sui mercati dei tassi di interesse fa capire che non è che qualcuno ci guadagna e altri no: il mercato alla fine è lo stesso; i consumi scendono giù in tutti i Paesi

luogo nel quale tutti dovranno dire la loro sulla questione del lavoro, perché è da lì che si parte. E ovviamente, ognuno la dovrà declinare a suo modo. C'è chi dovrà parlare delle proprie deficienze nazionali. Maria Grazia Gatti ha fatto riferimento ai servizi all'impiego: riprendo questo punto perché è chiaramente uno dei nostri principali problemi,

Ancora, il collega De Cristofaro ha parlato della questione dei paradisi fiscali, tema del quale il Consiglio europeo del 22 maggio ha discusso, arrivando a conclusioni secondo me molto importanti.

dimenticata di tutte le politiche contro la scarsa attenzione che viene posta rispetto al tema della fedeltà fiscale)

sono rimasto molto colpito dall'atteggiamento della Presidenza britannica del G8: la Gran Bretagna è legata ad una serie di territori

che abbia conti correnti nei paradisi fiscali può immaginare che vi sia lo stesso clima di dieci anni fa, non è così: la pressione che oggi c'è e ci sarà

asimmetria tra chi paga tutte le tasse fino all'ultimo centesimo e chi invece toglie dall'attenzione della comunità dalla partecipazione alle spese comuni

fiscalizzati rappresenta uno degli elementi attorno ai quali essa costruisce tutto ciò che di negativo anche nel nostro Paese su questi temi avviene. Ho citato questi temi perché il Consiglio europeo del 22 maggio

stanno facendo vivere situazioni drammatiche a parti crescenti delle nostre popolazioni. Attorno al tema della lotta alla povertà

chi è in condizioni di povertà estrema spesso e volentieri non è cittadino dell'arena politica: spesso e volentieri nemmeno partecipa, né vota, non è organizzato e, quindi, non è in grado di far valere la sua voce e di ottenere spostamento di risorse e di attenzione attorno a suoi bisogni che non vengono dal circuito elettorale considerati come utili e fondamentali. passo in questa direzione. Considero però molto importante che questo tema abbia fatto capolino nel corso della nostra discussione di oggi, perché è parte integrante del ragionamento che cercheremo di portare nel dibattito europeo. Molti interventi hanno fatto riferimento alla questione della costruzione europea e - riprendo un passaggio del senatore Volpi - dell'anima da rimettere dentro la costruzione europea. Credo

la politica torna a guidarla. un riferimento alla distinzione fondamentale tra politica e politiche (che rimane una distinzione, secondo me, di saggezza nella situazione politica particolare che il nostro Paese sta vivendo), ritengo però che quella europea sia una vicenda in cui - concordo - o c'è guida politica, visione politica e il senso da parte di ognuno di noi di una missione politica, oppure non c'è nessuna possibilità di farcela. L'Europa non crescerà

scaricare la nostra frustrazione contro gli eurocrati o contro tutto ciò che di tecnocratico ci può essere a Bruxelles: il problema siamo noi che lasciamo quello spazio.

per la politica, e nelle scelte che dobbiamo fare, e nel capire che attorno a queste scelte bisogna fare delle modifiche coraggiose. Giorgio Santini ha fatto riferimento alla questione dei fondi strutturali. Vogliamo continuare ad essere il Paese che spende peggio i fondi strutturali? È colpa di qualche eurocrate di Bruxelles se noi spendiamo male i fondi strutturali, o non è forse colpa nostra

...*alla vicenda europea che tornano indietro a noi come fondi strutturali e che noi regaliamo al Portogallo e all'Irlanda perché li usano meglio di noi. È giusto questo? È colpa di qualcuno a Bruxelles? No, è colpa nostra. Vorrei che questa fosse la consapevolezza profonda con la quale, attorno a tutti questi temi, cerchiamo di andare avanti. Voglio concludere riprendendo l'intervento del senatore Carraro,

Siccome penso anche io che sia uno scandalo, che ci siano, non soltanto nelle società private ma nelle società pubbliche dirigenti che guadagnano multipli assolutamente insopportabili rispetto a quello che guadagna un qualunque dipendente pubblico... Oggi mi sento anche un pochino più tranquillo perché, come sapete, avendo il Governo sui propri stipendi fatto una scelta e cioè avendo eliminato lo stipendio da Ministro e da Presidente e mantenuto solamente unico stipendio quello da parlamentare, per me sarà più facile andare a parlare con alcuni *manager* pubblici e dire loro: «Non credo sia giusto che tu guadagni 30 volte quello che guadagna il Presidente del Consiglio del tuo Paese che ti sta nominando»

lo dico perché troppe volte anch'io sento ripetere: «Il 3 per cento... ma in fondo la Francia e la Spagna... Perché non anche noi? Così abbiamo qualche soldo in più». Voglio insistere su questo punto. Per noi, oggi, uscire dalla procedura di infrazione vuol dire È come nel ciclismo.

è la più difficile: abbiamo il gran premio della montagna, adesso. La seconda fase: avremo il falsopiano a fine anno. La terza fase: avremo la discesa nel 2014. Perché cito questo? questo? Ovviamente oggi siamo in fase d'uscita dalla procedura di infrazione. L'uscita avverrà giovedì e venerdì, ed è evidente che la rigidità è dovuta al fatto che siamo in un bilancio 2013. Ed è un bilancio 2013 nel quale possiamo coprire ciò che vogliamo fare soltanto con coperture dentro il bilancio. È chiaro a tutti questo. Non abbiamo margini di flessibilità in più, perché il bilancio è quello di quest'anno,

un passo di pianura, perché io conto che saremo in grado di avere due risultati positivi. In merito al primo risultato positivo, si tratta dei primi risultati sul bilancio pubblico e sull'economia dell'operazione di immissione di quelle decine di miliardi di pagamenti dei crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione, che rappresenta e ha rappresentato negli anni scorsi una delle più grandi richieste che tutti noi abbiamo rivolto al nostro Stato, e che oggi è in corso di pagamento ed avrà effetti benefici sul bilancio pubblico, in termini di entrate fiscali (lo sappiamo, l'IVA), e speriamo naturalmente in termini anche di crescita dell'economia. oggi lo devo dire con più prudenza rispetto alla settimana scorsa: se continuasse una tenuta dei tassi di interesse sul nostro debito pubblico, saremo in grado alla fine dell'anno di avere un po' meno peso sulla cifra complessiva annuale del nostro servizio sul debito, che ovviamente dipende tutta da quel livello dei tassi di interesse. Questo vuol dire avere alla fine dell'anno la pianura. Poi l'anno prossimo, la discesa. Certo, non sarà una discesa in picchiata, ma alle volte è anche meglio avere una discesa un po' più piana per evitare di farsi del male. Quindi, sarà una discesa, e lo sarà perché potremo gestirci grazie all'essere usciti dalla procedura con maggiore flessibilità. Con il bilancio 2014 che faremo in questa sede - il Governo lo proporrà e il Parlamento lo discuterà, lo cambierà e lo approverà nella legge di stabilità che faremo insieme nell'autunno di quest'anno - saremo in grado di usare quella flessibilità che quest'anno più di tanto non siamo in grado di usare, perché non saremo più il sorvegliato speciale. Il bilancio ce lo faremo noi. Non saremo più nella procedura, perché la procedura non è un fatto solo politico ma anche giuridico e formale. Non essere più lì dentro vuol dire avere un margine di lavoro che ci consentirà di scegliere insieme. Ecco perché io dico che dobbiamo essere realisti, pragmatici, ma sono ottimista rispetto a questo percorso. Se faremo il gran premio della montagna adesso, se faremo la pianura poi, la discesa del 2014 ci consentirà di andare a guidare l'Europa nel secondo trimestre e fare, in quella sede, in quel momento, quel passo decisivo verso gli Stati Uniti d'Europa che - fatemelo dire con un po' di orgoglio nazionale - solo una Presidenza italiana dell'Unione europea sarà in grado di far fare all'Europa.

del Consiglio, anche a nome del Gruppo Per le Autonomie ribadisco la nostra piena sintonia con quanto da lei affermato, anche per l'approccio che ha avuto nei confronti Grazie, di quasi tutti coloro che oggi hanno parlato. Abbiamo apprezzato, in particolare, il linguaggio della verità e della realtà che lei ha adottato: da una parte, ha parlato dell'Europa vera, di quella fatta dalle imprese, dai giovani, dalle famiglie e dai territori; dall'altra, però, ha parlato anche di un'Europa che ha bisogno di visione politica, politica, di vivere anche di ideali e di coltivare la speranza. È un atteggiamento che finalmente guarda all'Europa secondo le regole di un rapporto giusto e nel rispetto da parte dell'Italia delle regole che l'Europa PANIZZA). Credo che questo sia anche il giusto approccio che dobbiamo avere per recuperare la fiducia anche degli altri Stati europei, e vorrei dire anche per la giusta dignità che il nostro Paese deve avere nei confronti dell'Unione.

la proposta di risoluzione n. 5 che racchiude peraltro tutte le componenti pratiche, le indicazioni e le direttive chiare che lei ha voluto anche oggi elencare.

l'impegno a promuovere il potenziamento della strumentazione e della dotazione finanziaria dell'Unione europea per sostenere l'economia, tutti i progetti volti a contrastare la disoccupazione giovanile, e in particolare il fondo a cui lei ha accennato in maniera molto chiara e dettagliata. E ancora, il collegamento tra le politiche attive del lavoro e il circuito scuola-università-lavoro, che è sempre stato al centro anche dell'interesse espresso dal nostro Gruppo; il riferimento all'unione bancaria e, quindi, alla necessità di creare regole bancarie che tutelino i risparmiatori

di finanza pubblica, il contenimento del debito pubblico, la volontà di dare attuazione ed effettività alle riforme già in atto, la promozione nel settore bancario delle pratiche di governo societario, le iniziative di riforma del mercato del lavoro, la riduzione della pressione fiscale (misura peraltro contenuta anche all'interno di una delle risoluzioni che oggi saranno, credo, approvate). E poi, il mercato nel settore dei servizi e, infine, la volontà di ridurre il numero delle infrazioni da parte italiana, per dimostrare che l'Italia crede nell'Europa e ne rispetta le regole. Ci fa, inoltre, piacere prendere atto risoluzione a fare in modo che il semestre di Presidenza italiana possa essere davvero un semestre costituente, che ci porti ad avere istituzioni europee più democratiche, trasparenti, efficaci ed efficienti. Le sue dichiarazioni di oggi ci fanno ben sperare e credo che ci avrà tutti al suo fianco nel momento in cui cercherà di restituire passione e credibilità all'Europa e di fare in modo che questa Unione sia davvero vicina ai territori, alla gente e alle imprese, che ne costituiscono la spina dorsale.

signor Presidente del Consiglio, il dibattito svolto dai politologi nel più recente passato ci ha abituati ad individuare la contrapposizione tra due modi di fare politica:

e di avere la responsabilità di trasferirla al vissuto sociale; dall'altra parte, l'idea che ormai la politica si sia trasformata in una modalità di svolgimento di tipo aconfessionale e che, quindi, il politico, per aver il maggior successo possibile, debba governare non già secondo la confessione posseduta, cioè secondo il suo ideale di società, ma secondo quello che interpreta essere il migliore desiderio dell'elettore e del popolo votante.

in atto sia da prendere in considerazione e non penso che nell'espressione del nostro voto dobbiamo fare riferimento a quello che riteniamo o crediamo il popolo voglia, bensì a quello che è il nostro convincimento.

dobbiamo azionare la nostra politica di sostegno e far sì che quella sia la politica del Governo. Tante volte ci troviamo nella difficoltà di convincere in tal senso i nostri amici ed elettori Tante volte, credo, il Governo si troverà nella difficoltà di convincere non amici, non Regioni, non politici, ma Stati interi che si producono in una politica di euroscetticismo.

ho detto che era ben strano che il Regno Unito partecipasse alle riunioni e che non avesse sottoscritto il Trattato sull'Unione monetaria. Il rappresentante del Parlamento britannico, in un modo molto sornione e molto inglese, mi disse di essere d'accordo con me, ma che, purtroppo, il suo accordo era condiviso soltanto dal suo gatto. Lei, signor si ritroverà nei prossimi giorni, non soltanto a dover convincere gli inglesi, ma dovrà prodursi in un'azione specifica per cercare di volgere al meglio l'interpretazione che dell'Europa e degli Stati Uniti d'Europa hanno avuto i colleghi germanici. E i colleghi germanici sono giustappunto, e giustamente, convinti di essere dalla parte della ragione quando finiscono per essere rispetto all'unione bancaria e all'unione fiscale

In quel caso, gli amici che rappresentano il Nord Italia non pensano che quelli sono soldi italiani, ma, visto che il 20 per cento dei tributi italiani viene pagato da un 10 per cento della popolazione (che sono gli abitanti della Lombardia), essi hanno giusta ragione di pensare che quei soldi siano soldi loro. Quando facciamo riferimento all'Europa, i colleghi germanici hanno tutti i buoni motivi di pensare che le risorse europee siano risorse loro, perché loro hanno un fatturato di circa 3.500 miliardi

mentre noi ne esportiamo 500 e, insieme alla Francia e alla Spagna, non raggiungiamo il monte di esportazioni dei tedeschi (perché raggiungiamo la cifra di 1.200 miliardi, contro, appunto, i 1.400 della sola Germania). La Germania, a questo punto, fa un ragionamento

del denominatore del rapporto *deficit*-PIL? Anche perché abbiamo visto che questo è ciò che, negli Stati Uniti d'America e in Giappone, non funziona più. Ella, nel suo intervento, pronunciato tre frasi sintomatiche in proposito. Le cito, perché le ho rilette: dobbiamo batterci contro una tendenza insidiosa all'inerzia, contro un'ostinata difesa di rigide impostazioni e contro una protezione egoistica di prerogative nazionali. Credo che lei oggi deve ricevere, come Governo, il nostro incoraggiamento, perché il contrasto, che la politica italiana deve avere rispetto a chi ha una tendenza insidiosa, una posizione egoistica e una ostinata difesa deve essere supportato e ben difeso dal voto del Parlamento.

parlamentare e rappresentante di una piccola parte politica, che i tedeschi hanno cominciato le loro contrapposizioni mondiali da sicuri vincitori, e poi hanno perso sempre le guerre. Questo bisogna ricordarlo a loro e anche a noi, perché noi dobbiamo dobbiamo essere confessionali a tal proposito e dobbiamo produrci in un'azione di contrasto che, passo dopo passo, ci conduca all'unione all'unione politica. Da questo punto di vista (il passo dopo passo), quando il 27 e il 28 giugno sarà in discussione l'unione bancaria, mentre il voto sull'unione bancaria è un'azione che ha difficoltà ad essere letta da quell'elettore che dobbiamo convincere per le nostre buone ragioni, dobbiamo parlare di ciò di cui ella sta parlando: del fatto, cioè, che, contemporaneamente all'unione bancaria, di difficile lettura, noi ci si produca in una attenta politica per i giovani. la prima ci porterà all'unione fiscale ed economica, la seconda rappresenta il primo passo per arrivare all'unione politica.

è cosa diversa dal consumismo. Nel secolo scorso, i migliori periodi si sono avuti quando c'è stato il consumo, non il consumismo. I critici del *New Deal*

Solo se stimoliamo l'avvicendamento generazionale possiamo garantire questo e sperare che il vecchio continente diventi un nuovo continente.

la più drammatica delle emergenze da quando ha avuto inizio la crisi. Una crisi che molti, per troppo tempo, si sono illusi riguardasse solo la finanza. Troppo tardi ci si è resi conto dell'entità e della natura di un fenomeno che colpiva le economie più avanzate, provocando effetti più prolungati nel tempo di quanto si sia mai visto dal dopoguerra ad oggi. Soprattutto, in Europa, abbiamo colpevolmente lasciato che questa crisi agisse in profondità per molto tempo, ancora di chiamarla con il suo nome; che distruggesse capacità produttiva, lavoro, competenze, prima di accorgerci che c'era bisogno di risposte e soluzioni non scontate. Le istituzioni europee - e questo è per noi uno dei punti decisivi - hanno una parte di responsabilità che riguarda la gestione di questa crisi. In Europa abbiamo sentito ripetere che si trattava di crisi dei debiti sovrani, cioè dei singoli Paesi. E ci è stato spiegato, sempre dagli organismi europei, che il tempo degli sprechi era finito, che alla gestione dissennata delle finanze pubbliche fosse dovuta la ricaduta più pesante degli effetti della crisi e che l'austerità fosse l'unica cura praticabile, dura ma inevitabile. Eppure, onorevoli colleghi senatori, i conti non tornano. Applicando quella cura gli effetti della crisi si sono approfonditi, le difficoltà delle economie nazionali sono aumentate, i redditi sono precipitati verso il basso, la coesione sociale ha iniziato a soffrire come mai avvenuto da decenni. Ne abbiamo sotto gli occhi gli effetti drammatici in Grecia, in Portogallo, in Spagna. Questi Paesi, dopo la cura, non stanno affatto bene; ma neanche noi siamo molto in salute. Non penso che dire questo significhi essere antieuropeisti. Dire che l'austerità sta uccidendo il sogno dell'Europa significa, al contrario, assumersi una responsabilità politica verso l'Europa. Chi come noi crede che il nostro futuro debba essere quello degli Stati Uniti d'Europa pensa che questo continente non può essere agli occhi dei suoi popoli soltanto istituzioni che smantellano i diritti in nome di una ripresa che si allontana sempre di più e che proprio per questo, richiede sacrifici sempre più grandi. I risultati li abbiamo davanti agli occhi guardando soltanto alla stato del nostro Paese. Dopo la robusta cura di austerità praticata dal Governo Monti, il PIL ha registrato un segno negativo e la disoccupazione è aumentata, senza tenere nemmeno conto della cassa integrazione e della disoccupazione sommersa. Si tratta della fotografia di un Paese in sofferenza, al punto di veder sprofondare il suo comparto produttivo. Dal 2008, l'economia ha visto dissolversi circa il 25 per cento delle sue capacità, mentre sull'occupazione gli effetti sono stati drammatici: ne abbiamo parlato in precedenza e non c'è bisogno di aggiungere altro. Va da sé, appunto, che i soggetti più deboli siano quelli che hanno pagato di più il prezzo della crisi e delle politiche sbagliate. I numeri drammatici sono abbastanza per per parlare, in relazione alle giovani generazioni, di una vera e propria generazione perduta. Dunque apprezziamo l'impegno dei Paesi europei: purtroppo, però, questo dispendio di energie, anche comunicative, a nostro avviso ha prodotto un risultato ancora insufficiente se in definitiva parliamo, come sembra, tutt'al più dell'anticipo del fondo operativo per l'occupazione giovanile, che arriverebbe ad una somma troppo modesta, divisa per di più tra il 2014 e il 2015, e comunque senza nemmeno un accordo comune su questa misura. Tuttavia, è comprensibile che oltre un certo limite, peraltro risicato, non si possa andare ed è proprio questo il punto. Capiamo bene perché sia bastato ipotizzare il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti o chiamare in causa la Banca europea per gli investimenti per aggirare il *credit crunch,* che paralizza l'economia e mette fuori gioco piccole e medie imprese, che a stretto giro si è avuta la risposta dei guardiani dell'austerità. una risposta che non promette nulla di buono e allontana anche solo l'ipotesi della *golden rule*, che permetterebbe di scomputare gli investimenti dal calcolo del *deficit* di bilancio, caricando cioè tutto il peso politico in direzione dell'unione bancaria e senza troppo concedere alle questioni sociali sul tappeto. Evidentemente una boccata d'ossigeno non è consentita a chi sta morendo strangolato dall'austerità.

per sottacere che le riforme strutturali che il Consiglio europeo chiederà di portare avanti nelle sue conclusioni sono troppo simili a quelle che hanno reso difficile mettere in campo anche quelle politiche attive per l'occupazione, su cui pure il Consiglio ha deciso di lavorare. Riteniamo viceversa che anche per la realizzazione della vera unione politica del continente sia necessario e indispensabile rompere la gabbia dell'austerità, a partire dalla radicale modifica del trattato sulla convergenza dei bilanci, ovvero il *fiscal compact*, di cui abbiamo già parlato, che riteniamo una delle cause delle difficoltà. Pensiamo cioè che vada stabilita una priorità degli investimenti nell'economia reale, a partire dal rilancio del mercato interno, tramite una politica di redistribuzione dei redditi che favorisca la domanda, anche attraverso una trasformazione del modello di sviluppo. modo riteniamo - e ci associamo a chi lo ha detto - che sia indispensabile lavorare sin da subito alla costruzione di un sistema continentale di reddito di cittadinanza. Come ha scritto Ulrich Beck - che lei, signor Presidente, conosce bene - un grande intellettuale europeo prima ancora che tedesco (se posso dire così): «Ci sono i tempi della piccola politica di esecuzione delle regole, e c'è un tempo per la grande politica di cambiamento delle regole». Noi pensiamo che non sia più il tempo della piccola politica, ma che sia arrivato il tempo in cui l'Unione europea metta mano ad una grande politica di cambiamento delle regole dell'austerità, che stanno appunto distruggendo il sogno europeo e che stanno seminando paura e divisioni tra i suoi popoli. Un nuovo programma europeo, un *social compact* - lo vogliamo chiamare così - vincolante per gli Stati, che finalmente parli di sviluppo sostenibile, di coesione sociale, di lotta alle disuguaglianze e di lotta alla povertà.

A questo Consiglio europeo la stampa e le istituzioni dedicano una grande attenzione. Penso che l'importanza vada riconosciuta ai temi sul tavolo, in particolare a quello dell'occupazione o, più giustamente, della disoccupazione, soprattutto quella giovanile, come lei ha ricordato. Che il tema sia urgente e inderogabile è fuori discussione, Che il Consiglio europeo sarà adeguatamente decisivo e risolutivo a tal proposito è invece poco credibile. Nel nostro Paese, nel primo trimestre del 2013, il tasso di disoccupazione è salito al massimo storico dal 1977: siamo ad oltre il 12 per cento. Ma il dato più preoccupante riguarda la disoccupazione giovanile. Come ricordato, tra i 14 e i 25 anni siamo ad oltre il 40

presidente Letta, è che la pressione fiscale si attesta al 53 per cento, è tra le più alte del mondo, e la pressione reale, che è quella che interessa alle nostre imprese, per cento, tanto che i nostri artigiani lavorano per lo Stato fino a settembre, tenendo per sé e la loro famiglia solo quello che rimane negli ultimi quattro mesi.

rispetto alla tassazione che c'è in Italia, possiamo tutti considerarla un paradiso fiscale. Il costo del lavoro è diventato intollerabile per le aziende ed anche per i lavoratori; occorrono risorse per interventi di riduzione, attraverso una detassazione e una decontribuzione a carico dei datori di lavoro; bisogna ridurre il cuneo fiscale. Solo così sarà possibile dare alle imprese una boccata d'ossigeno e potenziarne la competitività, creando creando un circolo virtuoso impresa-economia-occupazione. Servono anche politiche di flessibilità del mondo del lavoro; dobbiamo coniugare le esigenze sentite dalle aziende con la certezza del posto di lavoro richiesta dai giovani, e dai meno giovani, inoccupati o disoccupati.

Questi non sono dati che sono venuti alla luce in una notte; eppure solo oggi, dopo sei anni di crisi economica, il massimo organo comunitario dice che la priorità della propria azione di intervento deve essere il lavoro, senza peraltro arrivare a riconoscere chiaramente quanta di questa crisi sia stata addirittura provocata dalle politiche sbagliate imposte dalla stessa Unione europea agli Stati membri. Porre con così grave ritardo la questione della disoccupazione come punto qualificante dell'agenda europea è già di per sé la più chiara attestazione del fallimento profondo del percorso comunitario. E purtroppo sappiamo anche già che il prossimo Consiglio europeo, secondo un rituale che ormai conosciamo, sarà una riunione di Capi di Stato e di Governo, le massime rappresentanze istituzionali, che in diverse pose si presteranno a foto ricordo, a strette di mano, con o senza cravatta, a *flash* e a riprese dei *media*, prima e dopo aver firmato un documento conclusivo del vertice, l'ennesimo, fatto solo di linee programmatiche e formule di rito. Questo appuntamento di giugno, che dovrebbe servire ad un confronto tra i Paesi membri, per coordinare e decidere insieme le politiche economiche, è diventato il momento in cui i rappresentanti europei eletti dal popolo ratificano senza colpo ferire i *diktat* della Commissione europea. Il Consiglio è ormai niente più che un megafono delle ricette deleterie di un gruppo di burocrati, particolarmente rigidi e inflessibili con alcuni Paesi, quelli più deboli e in difficoltà, e più accondiscendenti con chi rappresenta il maggiore potere economico e finanziario del territorio europeo. Sul nostro Paese, tanto per fare un esempio, il Consiglio europeo ci ricorderà che la Commissione ha acconsentito a chiudere la procedura di disavanzo eccessivo, senza che peraltro ciò comporti concretamente alcun sospiro di sollievo per la nostra economia, salvo evitare ulteriori assurde sanzioni che proprio l'Esecutivo comunitario avrebbe potuto imporre. Il Consiglio europeo proporrà, con il plauso del Governo italiano, l'ennesima strategia per la crescita e la lotta contro la disoccupazione, riproponendo formule cariche certamente di buone intenzioni ma di scarso valore concreto. L'occupazione, caro Presidente, non si crea per legge; si crea in un sistema economico dinamico, produttivo, favorevole alle imprese, funzionale, e in un mercato fatto di persone che guardano al futuro con fiducia. Quello che la Lega propone, anche con il documento che sottopone al voto, è un cambio di passo, ma un cambio di passo vero. Le politiche comunitarie che abbiamo fin qui conosciuto, questa macchina europea, hanno dimostrato tutta la loro debolezza, inadeguatezza e rigidità. Così non si può andare avanti. Nulla potrà fare l'Unione europea contro la crisi economica, che sta distruggendo decenni di sviluppo industriale e sociale, se non partendo da una profonda e totale rivoluzione di se stessa. L'Europa, come contenitore di mere politiche economiche o commerciali, oggi non solo non serve più, ma è diventata quasi un ostacolo e sicuramente un bersaglio del malcontento sociale e popolare. Pena la sopravvivenza della stessa idea d'Europa, oggi i cittadini europei non guardano più all'Unione europea con la fiducia con cui si guarda a un progetto, ad un sogno, a un ideale di pace e di benessere (per il quale è nata), ma si guarda a Bruxelles con il timore di un tutore troppo sordo e severo, che i popoli europei non amano e a cui non credono, che non vuole il nostro bene, ma guarda solo a concetti sterili: il rigore di bilancio, la stabilità dei prezzi, indipendentemente dalle condizioni di vita delle persone. *(Applausi dal Gruppo* di reagire e gestire il grave momento attuale è andata di pari passo con l'imposizione a molti Paesi di misure economiche draconiane, impedendo quindi sul fronte interno qualunque possibilità di intervento a sostegno delle economie nazionali e locali. Nel nostro Paese ne abbiamo avuto un assaggio con la famosa lettera della BCE dell'autunno 2011, che ha addirittura determinato la fine di un Governo e l'avvio del commissariamento forzato da parte di un Esecutivo di tecnici. Oggi sappiamo che quel Governo, concepito dai salotti europei, ha fatto tanti danni e nessuna riforma decisiva,

che ormai, però, ha già distrutto in maniera irrimediabile il mercato immobiliare edilizio bloccando i consumi delle famiglie; deve congelare l'aumento dell'IVA, che colpirà pesantemente le famiglie e i consumi. Signor Presidente, non prendiamo in giro gli italiani. Un rinvio di tre mesi non serve a nulla. Non nascondete la polvere sotto il tappeto: non serve. I risultati dannosi delle politiche perseguite dalle autorità europee, con la complicità delle altre organizzazioni internazionali, a partire dal Fondo monetario internazionale, nei confronti dei Paesi in condizioni di maggiore difficoltà, sono ormai palesi ed esplicitamente contestati addirittura da alcuni degli stessi responsabili. Esempi a riguardo appaiono le autocritiche del Fondo monetario internazionale nei confronti della strategia drammaticamente recessiva adottata per la Grecia, così come gli assurdi sacrifici imposti ai risparmiatori di Cipro. Proprio quella autorevolezza e quella credibilità che un organismo come l'Unione europea doveva offrire ai suoi Stati membri per rafforzarsi sulla scena internazionale sono state distrutte dalle scelte della *troika*, imposte violando la sovranità dei Governi eletti e le promesse fatte in passato. in grado di rispondere efficacemente alle urgenze determinate dalla crisi economica, occupazionale e sociale, avviando subito una profonda revisione dell'architettura istituzionale europea, volta alla realizzazione dell'unione politica federale, sulla base degli esiti di una consultazione popolare referendaria che coinvolga tutti i popoli europei.

desidero esprimere al presidente Letta i rallegramenti di Scelta Civica, nonché quelli calorosi che gli rivolgo come suo predecessore nella guida del Governo. Ringrazio lei, signor Presidente, e quanti in altri interventi hanno, come lei, voluto sottolineare elementi di continuità tra l'azione del precedente Governo e di quello da lei presieduto. Non sarò quindi io a mettere in luce l'aspetto della continuità, se non quello che ascrivo a suo merito, signor Presidente, di una visione strategica del rapporto tra l'Italia e l'Unione europea, che fa parte della sua cultura come della nostra, come già ha posto bene in luce il senatore Casini. All'interno di questa comune visione strategica vi è un aspetto, questo sì, che voglio sottolineare. Lei e noi abbiamo in comune la rivendicazione di un ruolo forte, non subalterno, dell'Italia in Europa; un ruolo da protagonista dell'Europa, non da antagonista dell'Europa o di singoli Paesi ritenuti guida dell'Europa. Tuttavia, per essere protagonisti occorre non trovarsi in condizioni di debolezza, non essere sorvegliati speciali, non dipendere dalla benevolenza altrui. Lei, signor Presidente, ne sono certo, farà buon uso, con l'autorevolezza che in pochissimo tempo si è già conquistato in quei circuiti e nell'interesse dell'Italia, dello spazio di autonomia che il nostro Governo, con l'appoggio del Parlamento, nella precedente legislatura ha teso a riconquistare per l'Italia. quello che lei prospetta come azione del Governo, quello che il Parlamento la incoraggia a conseguire in Italia e in Europa, non sarebbe possibile; a dispetto delle sue qualità personali, lei non avrebbe l'autorità politica e nazionale per farlo, farlo, se giovedì e venerdì sedesse al Consiglio europeo come titolare di un Paese gravato non soltanto da un altissimo debito, ma da una procedura di disavanzo eccessivo ancora in corso. Men che meno lei avrebbe potuto presentarsi con la sua dignità e con il peso dell'Italia a quel consesso se il suo predecessore avesse ceduto alla via facile, prudente, consigliabile, che in effetti ci veniva consigliata dalle autorità monetarie e finanziarie internazionali nonché da alcuni Governi d'Europa. In

La nostra risposta è sempre stata: perché non vogliamo che l'Italia perda sovranità in modo asimmetrico.

controreazione all'interno del Paese, a toni sempre più rancorosi, provinciali, irrealistici e impresentabili, se l'Italia avesse dovuto elemosinare. La *troika* a Roma non l'abbiamo voluta. ci veniva consigliato di chiedere alla *troika* di venire a Roma, anche perché qualche mese fa, prima delle elezioni, c'era molta sfiducia che erroneamente serpeggiava negli ambienti internazionali; allora noi dicevamo che le elezioni ci sono in ogni Paese e chiedevamo perché si temevano

Non è questa l'Italia che vogliamo, ma è stato necessario fare un duro lavoro, con l'appoggio del Parlamento più o meno convinto, a seconda dei singoli provvedimenti, e con l'appoggio grande del Paese, che non ci sarebbe stato (ne sono convinto, anche come relativa tranquillità sociale, pure in una fase di grande pena e sofferenza) se quei sacrifici fossero stati visti come imposti da tecnocrati, quelli sì, nella nostra capitale e facenti parte di un'istituzione, magari di oltre Atlantico, che un anno dopo avrebbe pubblicato una nota per spiegare che aveva fatto grandi errori. Noi a questo ci siamo sottratti, e confesso che, solo vedendo lei in quella posizione, sono convinto che abbiamo fatto una buona cosa, perché della libertà che così l'Italia ha mantenuto, e anzi accresciuto, lei farà buon uso. Presidente, lei ha usato le espressioni «confronto duro», «confronto su basi politiche». Sono sicuro che saprà anche avere confronti duri. Credo che dobbiamo tutti smettere di pensare che le posizioni della Germania siano assurde e non siano modificabili con il convincimento. Le posizioni della Germania possono essere estreme su singoli aspetti, ma non sono assurde: avessimo avuto prima il Trattato di Maastricht e il Patto di stabilità, non avremmo creato la disoccupazione giovanile che c'è oggi in Italia, che attribuiamo all'Europa anziché ad una costruzione troppo tardiva dell'Europa, mentre per decenni in quest'Aula e in quella di Montecitorio si sono fabbricati volumi enormi di debito pubblico, che si diceva (gli economisti, non l'opinione pubblica) si sarebbero tradotti in un aggravio per le generazioni future. Le generazioni future sono arrivate e sono i nostri giovani disoccupati. le posizioni della Germania - lei lo sa, ha avuto gli incontri necessari a questo scopo ‑ possono essere oggetto di ragionamento, di analisi e di critica. Lei ha avuto la gentilezza, signor Presidente, di ricordare il contributo italiano al Consiglio europeo del giugno 2012 con

né doveva ricordarlo - uno strumento che le suggerirei magari di tenere presente nello sfondo della sua mente per uso raro ma incisivo: il veto costruttivo. La vera novità di quel Consiglio europeo non è stato il Patto per la crescita, ma l'aver ottenuto il meccanismo dello scudo *antispread*, com'è stato definito, oggi contestato - credo erroneamente - in Germania di fronte alla Corte costituzionale. quel caso ha dovuto fare uso del veto. Pur essendo tutti i 27, l'Italia *in primis*, a favore del Patto per la crescita,

dopo una notte di lavoro, anche la Germania ha modificato la sua posizione e quell'accordo c'è stato: non è stato la panacea, ma è stato l'ombrello intellettuale e politico che qualche qualche settimana dopo ha permesso al Presidente della Banca centrale europea di mettere in opera quello strumento, che peraltro l'Italia non ha voluto utilizzare perché non ve ne era bisogno e perché volevamo preservare intatta la libertà del futuro Parlamento e del futuro Governo.

la disoccupazione è drammatica, ma non credo si possa veramente ritenere che la responsabilità primaria di questo sia dell'Europa

su proposta di vari Governi, per tutelare sempre di più gli inclusi nei mercati, nelle professioni e nel mercato del lavoro, a danno degli esclusi e, in primo luogo, tale motivo, presidente Letta, se lei avesse la bacchetta magica e potesse tornare venerdì da Bruxelles avendo ottenuto l'abrogazione o la sospensione del Trattato di Maastricht e del Patto di stabilità, credo sarebbe una pessima notizia per l'Italia, oltre ad essere irrealistico. però, otterrà quanto occorre per dare un'intonazione più orientata alla crescita ed alle politiche europee. Lei dispone nel Paese di una grande coalizione che serve per sbloccare l'Italia attuando riforme che politicamente costano: si possono perdere le elezioni, ma cosa importa? una grande coalizione nata per sbloccare il Paese diventasse una grande «collusione» per frenare le riforme nel Paese, lasciando che prevalgano gli interessi... Presidente, inchinandomi anch'io alla memoria di Emilio Colombo: la sua storia di grande italiano costruttore d'Europa deve darci fiducia. L'Italia è stata fattore di impulso decisivo in tre momenti chiave: la decisione dell'elezione del Parlamento europeo a suffragio diretto (Parlamento che poi è stato presieduto proprio da Emilio Colombo);

sorretti in modo diverso da due grandi impegni nazionali, da due grandi coalizioni, avranno dato alla politica economico-sociale dell'Europa, anche con vantaggio per l'Italia, un assetto più equilibrato e più efficace nella *governance*, e intanto avranno modernizzato il Paese.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio dei ministri, colleghi, la strategia Europa 2020 si prefigge l'obiettivo di rilanciare l'economia degli Stati europei nel prossimo decennio, puntando su un'economia intelligente, sostenibile e solidale. L'Italia si dovrà dunque impegnare per il raggiungimento di tali obiettivi. Negli ultimi anni, il nostro Paese ha assistito alla crescita esponenziale del tasso di disoccupazione che, secondo l'ultimo rapporto ISTAT, è passato dal 6,1 per cento al 12,8 per cento del primo trimestre del 2013. Dal rapporto ISTAT dell'aprile 2013, risulta che i principali indicatori segnalano negli ultimi cinque anni evidenti difficoltà nell'ingresso e nella permanenza nel mondo del lavoro dei cittadini italiani. La crescita del tasso di disoccupazione è stata accompagnata non solo dalla perdita di occupati, ma anche dall'aumento delle forze lavoro potenziali, cioè inespresse (i cosiddetti inattivi), e dei disoccupati *part-time*. Chi sono le forze lavoro potenziali? Si tratta di cittadini che hanno perso la speranza di trovare lavoro o che non riescono nella loro ricerca. Quanti sono? Secondo gli ultimi dati ISTAT, sono più di 3 milioni i cittadini disponibili a lavorare o in cerca di lavoro e circa 3 milioni quelli che non cercano più lavoro che, sommati ai 3,276 milioni di disoccupati ed ai 605.000 sottoccupati, costituiscono un dato allarmante. Sono quasi 10 milioni i cittadini italiani che non percepiscono alcun reddito e che, quindi, sono a rischio di povertà e di esclusione sociale.

quasi il triplo della media dell'Unione. Si potrebbe cambiare l'articolo 1 della Costituzione, signor Presidente, nel seguente: «L'Italia è una Repubblica fondata sulla disoccupazione» Il nostro Paese è l'unico in Europa ad avere un così alto tasso di inattivi. In particolare, in Italia si trova un terzo degli 8,8 milioni di individui che nei Paesi dell'Unione europea dichiarano di non cercare lavoro.

I cittadini inattivi e disoccupati tra i 30 e i 54 anni potrebbero divenire un grave peso sociale per la nostra Nazione, in quanto privi di futuro, in totale rapporto di dipendenza nei confronti della previdenza sociale sono cittadini che non avranno modo di contribuire alla crescita del Paese dal punto di vista sia lavorativo che della crescita demografica; cittadini che non si potranno permettere di avere una famiglia. È una voragine del sistema economico e sociale del nostro Paese che non consentirà ad intere generazioni la progettualità del proprio futuro e la sostenibilità del proprio presente, con conseguente insostenibilità del sistema previdenziale. Chissà se i nostri Padri costituenti pensavano si potesse arrivare a questo! Un altro dato rilevante ed estremamente significativo è rappresentato dal progressivo aumento del peso economico degli ammortizzatori sociali. Dalla relazione dell'ISTAT si evince una caduta, una flessione dell'occupazione sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi in tutti i settori, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia, dell'industria e dell'agricoltura. Ciò ha portato all'impoverimento del tessuto produttivo italiano, all'incremento della disoccupazione con conseguente prevedibile futuro aumento degli stanziamenti di somme a favore del sostegno al reddito, e ad un aumento di cittadini che vivranno al di sotto della soglia di povertà. Non a caso il settore manifatturiero in Italia è in forte crisi e necessita di interventi sia immediati che a lungo termine. Sono 141 le vertenze industriali sul tavolo del Ministero dello sviluppo economico: 141 aziende che invocano l'aiuto del Governo per non affogare nel mare della crisi economica e che cercano in tutti i modi di tutelare il posto di lavoro di 111.000 operai a rischio. Lo ripeto, 111.000. Aziende quali Indesit, Berco, Merck, Omsa, Alcoa, Vinyls (potremmo elencare centinaia di casi) affrontano una crisi che coinvolge drammaticamente migliaia di lavoratori e di famiglie italiane. La globalizzazione ha causato la trasformazione della struttura del commercio mondiale, implicando notevoli impatti negativi sull'economia italiana, giacché chi ci ha governato non ha saputo gestire il cambiamento. Dall'acciaio al tessile, passando per le telecomunicazioni, gli elettrodomestici e il settore minerario: tutte realtà lavorative che entro settembre necessitano di trovare una soluzione positiva che permetta loro di non chiudere i battenti o di non trasferirsi all'estero. E non sono affatto sufficienti i quasi 30 miliardi di sussidi ed incentivi che ogni anno lo Stato distribuisce al mondo delle imprese per aiutarle a riavviare la propria attività o concedere ad esse una momentanea boccata d'aria. Gli effetti della globalizzazione riguardano anche l'aggiudicazione degli appalti, compresi quelli di servizi, con emissioni di bandi da parte della pubblica amministrazione italiana. Uno dei casi da citare è quello del gruppo Dussmann, multinazionale specializzata nella fornitura globale di servizi integrati per l'industria, la sanità, la scuola e le forze armate, vincitrice al ribasso di diversi bandi emessi da pubbliche amministrazioni. In svariati casi la succitata società non ha potuto sostenere la corretta gestione del servizio nonché il mantenimento degli *standard* occupazionali riducendo, pertanto, fortemente gli organici e generando numerosi contenziosi. Questo non è un caso isolato. Si inserisce nel disastrato quadro lavorativo italiano costellato di crisi aziendali, di utilizzi distorti della cassa integrazione ed è ancora più preoccupante se si considerano le prospettive future. All'interno degli obiettivi per il 2020 è incluso il raggiungimento del tasso di occupazione al 75 per cento (67 per cento per l'Italia). Già questo dato si commenta da sé. Come è possibile raggiungere un simile risultato in assenza di un vero e proprio passaggio di consegne tra una generazione e l'altra? Su cosa dunque dovrebbe puntare l'Italia? Quali azioni consentirebbero al nostro Paese di contribuire con pari dignità economica e sociale alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'Unione europea? Ciascuno Stato membro deve poter contribuire con pari dignità sociale ed economica all'Unione europea nel rispetto delle proprie vocazioni e capacità commerciali. La valorizzazione di agricoltura, arte, biodiversità, cultura, musica, beni architettonici, del *made in Italy* della nostra terra, insieme al rispetto della giustizia intesa come lotta all'evasione fiscale, insomma la valorizzazione della nostra civiltà, con l'aiuto dell'innovazione, costituiscono la ricetta per rendere la nostra nazione parte integrante e proattiva dell'Unione europea, non una palla al piede, non una preoccupazione per Paesi che hanno saputo investire su un mercato globale, ma parte necessaria ed integrante dello stesso. Nell'attuazione delle politiche sociali e dell'occupazione, nello sviluppo di politiche efficaci a combattere la povertà e a fornire assistenza alle categorie a rischio di esclusione sociale, si deve tener conto di dati differenti rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea: l'alta percentuale di inoccupati e disoccupati tra i 30 e i 54 anni, l'alta percentuale di donne inattive e, non ultimo, l'alto tasso di evasione fiscale. È necessario implementare un sistema virtuoso in cui il cittadino è al centro della vita della propria Nazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, un sistema di *welfare* che ponga fine alla frammentazione dei servizi per l'impiego dei programmi di politica attiva, l'istituzione di un unico osservatorio sul lavoro, il collegamento obbligatorio tra i Comuni, i centri per l'impiego pubblici e il sistema nazionale delle competenze certificate di ciascun cittadino. Un reale collegamento tra il sistema dell'istruzione e della formazione, l'istituzione del reddito di cittadinanza o meglio del reddito di dignità, già esistente nella quasi totalità dei Paesi dell'Unione, garantirebbero la flessibilità del mercato del lavoro, consentendo la formazione durante tutto l'arco della vita, la possibilità delle imprese di assumere i lavoratori reperendoli dal sistema nazionale unico delle competenze certificate ed ostacolando la progressiva marginalizzazione di chi ha la sola colpa di non poter più trovare lavoro in un Paese in agonia. La riduzione dell'orario di lavoro, poi, consentirebbe di creare nuovi posti di lavoro e la redistribuzione dei salari garantirebbe un sistema equo. È necessario intervenire in occasione del prossimo Consiglio europeo al fine di ottenere uno stanziamento straordinario di ulteriori risorse sia nell'ambito del Fondo sociale europeo per il finanziamento dei progetti volti a contrastare in maniera efficace la disoccupazione, sia nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Riguardo al Fondo di garanzia per i giovani, è indispensabile implementare azioni strettamente legate all'inserimento lavorativo del giovane. In tal senso, si deve porre in essere il superamento della cosiddetta staffetta generazionale

vuole uno Stato semplice, funzionale, così come l'avevano pensato i Padri costituenti, insomma efficace ed efficiente, uno Stato che rispetti la dignità del cittadino, che rimuova «gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Tutto questo si può raggiungere in un modo semplice: istituendo il reddito di cittadinanza.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, membri del Governo, colleghi senatori, nell'anticipare il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà

per avviare una politica finalmente mirata a quella che ella ha voluto definire crescita flessibile, ovvero alla chiusura della procedura per disavanzo eccessivo già accesa nei nostri confronti. Avvio della procedura - mi si consenta di dirlo - che si è poi rivelato un po' ingeneroso, se consideriamo il quadro generale di recessione e di conti in rosso nel resto d'Europa, e soprattutto se consideriamo le emergenze dei terremoti in Abruzzo e in Emilia-Romagna e in Emilia-Romagna che il Governo ha dovuto fronteggiare. L'Italia può indurre un forte stimolo verso una maggiore integrazione e deve avere se non l'orgoglio, la certa consapevolezza del suo *status* di grande Paese fondatore e di storico contribuente netto della comunità europea, nonché, ancora più importante, di seconda economia manifatturiera del continente. La crisi morde, lo sappiamo tutti, ma nessuno in Europa ora può veramente dirsene immune, nessuno può dire di possedere in esclusiva una ricetta vincente per combattere la recessione. Anzi, il prevalere finora di un rigore fondato soltanto sulla disciplina di bilancio ha indotto a scelte che si sono rivelate inappropriate e a misure incapienti, non adatte comunque alla gravità di una congiuntura che avrebbe dovuto imporre, soprattutto a chi è più forte e quindi chiamato a una *leadership* anche più coraggiosa, forse una maggiore lungimiranza. La lungimiranza e il coraggio sono ciò che dobbiamo chiedere ai nostri *partner*, ciò che ella sicuramente affermerà per il nostro Paese in occasione del Consiglio europeo, europeo, a cominciare dalla Germania, il cui orizzonte deve essere certamente più ampio e più prospettico delle proprie scadenze elettorali, che non possono certo orientare le nostre politiche domestiche, né tanto meno quelle Per riprendere le parole del senatore Monti, la Germania non deve essere neppure avara nell'aprire alcuni ombrelli intellettuali in fatto di crescita e occupazione e di quello sviluppo che è tanto importante, quanto consustanziale all'esistenza dell'Europa stessa. L'Italia, nonostante un debito pubblico purtroppo da primato (negativo) che deriva anche da una lontana eredità politico-amministrativa, rientra oggi nel ristretto numero di Paesi virtuosi dell'Eurozona (6 su 17), in linea con il vincolo del pareggio di bilancio già nel 2013. Un vincolo che il Governo e il Parlamento italiani hanno voluto addirittura inserire direttamente in Costituzione, dando anticipatamente corpo e sostanza alla nota *golden rule* europea. Da nessuna capitale, dunque, neanche da Berlino, c'è chi possa oggi rimproverare a noi di non esserci impegnati senza risparmio, di non aver compiuto sacrifici, di non aver fatto ciò che era possibile per rientrare nei faticosi e a tratti accidentati binari europei, anche a scapito - diciamocelo - dei nostri consumi e della nostra produttività. Semmai, gli errori nell'adozione di una politica troppo rigorosa sono stati indotti dal blocco dei Paesi settentrionali, in un contesto europeo non ancora davvero federale. L'Italia per prima, con Silvio Berlusconi presidente del Consiglio, già negli anni precedenti la crisi e, a maggior ragione, dopo che questa si è dispiegata in tutta la sua vastità ha segnalato all'Europa la necessità di un'interpretazione flessibile, intelligente, *ongoing*, continuativa, dei Trattati, che tenesse conto soprattutto dei cosiddetti fattori rilevanti, tra cui eventi eccezionali, crisi di significativa entità, debito aggregato, riforme strutturali attuate dai singoli Paesi. Questo certamente non significa per noi rinnegare gli accordi stipulati, né tanto meno volerli mutare *pro domo nostra*. Significa altresì attribuire, di volta in volta, alle specificità di contesto, alle disposizioni percettive, che calano nei singoli ordinamenti degli Stati membri, la funzione di equi adattatori di sistema, orientati all'economia e allo sviluppo comuni. Il Patto di stabilità era, ed è, un patto per la stabilità e per la crescita. E quest'ultima parte non la possiamo dimenticare mai. Per l'Italia questo è tanto più essenziale, direi vitale, in quanto il tessuto produttivo è costituito non già da multinazionali, da giganti economici, ma da qualcosa di molto significativo che è stato prototipo, ed è modello, formula studiata in tutto il mondo: una vastissima rete capillare, familiare, dinamica, costellata in una miriade di piccole, anzi micropiccole e medie imprese, che combattono contro una pressione fiscale spropositata e distruttiva, contro un costo esagerato dell'energia, contro lo svantaggio competitivo di una giustizia tardiva e quindi negata,

anche se noi li abbiamo purtroppo in larga misura in regime di monopolio, e che non possono essere risolti solo guardando all'Italia. Per questo noi crediamo nelle sue ferme intenzioni e confidiamo nelle indicazioni che impegnano il Governo a un confronto serrato, ad un negoziato assertivo con le istituzioni europee, al potenziamento di strumenti e quindi, per noi, alla realizzazione di riforme, che non saranno a costo zero, che svolgano una funzione anticiclica, ovvero espansiva, tali da mettere al centro le due assolute priorità che ella ha evidenziato: la ripresa della crescita e l'occupazione, anche e soprattutto giovanile. Il Gruppo PdL è pronto a sostenere il Governo nella richiesta di stanziare ulteriori risorse del Fondo sociale europeo contro la disoccupazione giovanile. È pronto a plaudire a una presa di posizione netta a Bruxelles per estendere le attuali opportunità di accesso al credito attraverso il Fondo di garanzia delle micropiccole e medie imprese; all'innesco di un processo riformatore della stessa *governance* europea, così come della Banca centrale europea, che dovrebbe avvicinarsi ai requisiti e alle prerogative di istituti centrali, che in Paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna e Giappone non solo tengono sotto controllo inflazione e prezzi, ma portano avanti coraggiose politiche procicliche per l'occupazione e la crescita e pratiche monetarie di ossigenazione dell'economia reale. Siamo d'accordo che per onorare gli impegni europei l'Italia dovrà proseguire in uno *screening* selettivo della spesa pubblica e soprattutto dare respiro alle famiglie perché riprendano a consumare, incrementando così la produttività e quindi vecchia e nuova occupazione. Ma la priorità delle priorità deve essere la drastica riduzione della pressione fiscale, da conseguire comprimendo la spesa pubblica improduttiva, i famigerati costi intermedi, e riducendo la voracità dello Stato anche nelle sue articolazioni territoriali. Siamo pure convinti che il semestre di Presidenza italiano dell'Unione europea nella seconda metà del 2014, che ella ha giustamente e anticipatamente (ma non troppo), ricordato possa e anzi debba essere contrassegnato come un semestre costituente, con l'ambizione di far procedere l'Italia e gli altri Paesi europei lungo un cammino complesso, che ha però

non hanno rappresentato la cura di un continente in crisi, ma ne hanno aggravato la malattia. Il PdL è infatti convinto che sia proprio questo il momento di dare una scossa all'Europa. Apprezzo la metafora del falso piano e della montagna. È tutto vero: *est modus in rebus*, e c'è il tempo per realizzare i singoli provvedimenti e i singoli progetti. Ma è ora che bisogna far ripartire l'Europa sulla base di un comune impegno al lavoro e alla crescita. Solo così, in fondo al *tunnel*, possiamo trovare quello che oggi sembra un miraggio abbastanza remoto: gli Stati Uniti d'Europa. Un miraggio, ma certo anche un esito suggestivo, perché l'Europa non può essere vaso di coccio tra giganti di ferro e trasformarsi, da grande sogno da realizzare, in obolo da pagare. Lo ripetiamo: basta rigore, basta austerità, o l'Europa muore. All'area storica di libero scambio è subentrata l'Unione monetaria, la *compliance* fiscale, e adesso, con qualche difficoltà, deve affermarsi l'unione bancaria. Ma come ci ricorda il presidente Letta il percorso è accidentato, anche perché qualche Stato *leader*, prigioniero di lacci congiunturali ed interessi localistici, mostra di non gradirla fino in fondo. L'Italia ha le carte in regola, ha le proposte giuste, ha l'umiltà ma anche la consapevolezza del proprio ruolo e, aggiungo, va a Bruxelles con un Presidente del Consiglio giovane, che conosce bene l'Europa, alla guida di un Governo che abbiamo voluto politico, non acquiescentemente tecnico, proprio perché fosse negoziatore forte dei nostri interessi e forte custode dei nostri diritti. Siamo certi che il presidente Letta lo rammenta bene: in Europa, con sé, avrà tutto il Paese. E, certamente, il nostro gruppo di parlamentari sarà a volte anche seriamente e costruttivamente critico verso questa Unione europea, ma sicuramente europeo

E su questi tre pilastri, che sono altrettanti impegni assunti davanti alle Camere, noi non potremo fare sconti. Presidente Letta, lei rappresenta tutto il Paese, un grande Paese, fiero del suo popolo, della sua cultura, della sua forza industriale, della sua inventiva imprenditoriale, della sua umanità, della sua volontà di riuscire. Con i nostri migliori auguri, Presidente, vada a Bruxelles, e ci faccia valere!

perché nel merito vi sono almeno tre aspetti molto importanti. Innanzitutto, il Consiglio europeo avrà al primo posto i temi dell'occupazione giovanile, come lei ha detto, e l'attuazione del patto per la crescita e l'occupazione, non proposti in contrasto con il risanamento necessario, ma con un profilo forte, visibile, più credibile rispetto a precedenti generiche affermazioni. Questo dato è un successo del Governo. Perché una svolta sui temi della crescita e dell'occupazione è premessa e condizione di altri traguardi, anche in chiave interna. È vero infatti che il lavoro lo creano le imprese e non le leggi, ma è altresì vero che senza l'impulso di politiche pubbliche mirate ed efficaci è difficile che le imprese ci provino; anche perché sui temi della crescita e dell'occupazione c'è pure una qualità da ricercare. La risoluzione lo dice, parlando di sostenibilità, innovazione, conoscenza, e noi siamo d'accordo. La proposta di risoluzione prende poi sul serio le raccomandazioni rivolte all'Italia dopo la chiusura della procedura di *deficit* eccessivo. È il secondo motivo del nostro voto positivo. Dobbiamo misurarci con le sfide lì contenute; il che non vuol dire accettare tutto passivamente senza svolgere un ruolo attivo. Oggi dobbiamo evitare due errori di segno opposto cui abbiamo assistito, ad esempio, ai tempi della difficile discussione sulla lettera della BCE, nell'estate di due anni fa. Da un lato considerare quelle indicazioni come dogmi, farle diventare tutta la nostra strategia, quasi fideisticamente. Dall'altro gridare all'ingerenza o cercare di sfuggire alle sfide e agli impegni che lo scenario europeo ci propone. Nessuna di queste due vie è feconda. Occorre accettare la prova, pur se ardua e di lungo periodo. Il tema del risanamento è in realtà nostro, non ci viene imposto da nessuno. E la nostra responsabile autonomia può esercitarsi su come l'obiettivo si raggiunge, sul *quantum* di equità, dì qualità, di coesione nazionale saremo capaci dì introdurre nelle manovre di aggiustamento budgetario. Tanto più chiaro e credibile sarà l'impegno a chiudere la stagione interminabile del debito, maggiore sarà lo spazio nostro per le esigenze di flessibilità e di adattamento alle nostre esigenze nazionali. Terzo punto chiave della proposta di risoluzione è la sollecitazione per una più forte Unione politica, sul terreno economico, fiscale e bancario e su quello della complessiva solidarietà istituzionale e politica. Senza ridurre questo pesante *deficit* di politica, di visione (come lei ci ha detto stasera), il compito nostro sarà molto difficile. È l'Europa il terreno dove si coglie meglio il nesso inscindibile fra sociale e istituzionale, tra economico e istituzionale. I cittadini chiedono interventi rapidi e incisivi, non possiamo rispondere solo con nuove architetture costituzionali, a meno che - e questo è il caso dell'Europa, lei lo ha detto - non risulti chiara la connessione tra riforma istituzionale e forte impatto delle misure economiche e sociali. Chi saprà spiegare e realizzare questo aggancio avrà un indubbio punto di vantaggio sul piano politico e su quello del consenso. L'Europa, presidente Letta, è il luogo dove si incontrano virtuosamente la «politica» e le «politiche», come lei ama dire. La politica intesa come visione, come progetto di futuro; le politiche viste come strumenti, come sistemi relazionali, come alleanze tra soggetti istituzionali e sociali. Due ultime riflessioni, signor Presidente, prima di chiudere. La prima è questa: la tematica europea dovrebbe appartenere alla ristretta cerchia del patrimonio condiviso dal Paese, dal suo ceto politico tutto, dal suo gruppo dirigente più vasto. Senza tema di esagerare, direi che dovrebbe stare, senza sfigurare, insieme alle regole costituzionali ed elettorali. Intendo in questo caso una generale accettazione della politica europeista, dei suoi valori e delle sue regole, ossia il quadro che definisce il «come» si opera, le regole dentro le quali ci si muove. Sul «cosa» fare, sulle scelte politiche e programmatiche, vale ovviamente il voto popolare, vale il principio di maggioranza così come organizzato nei Trattati dell'Unione. Oggi - e da qualche anno - c'è il segno della destra e del centrodestra sulle politiche europee, perché i partiti di destra e di centrodestra sono maggioritariamente prevalenti all'interno dei 27 Paesi membri e nel Parlamento europeo: è normale e giusto riconoscerlo e prenderne atto. In passato ci fu un segno diverso e così potrebbe essere anche in futuro. Tuttavia, consentire all'Europa di vivere e di pesare, anche prima delle sue scelte politiche e delle sue maggioranze, è tema che ci riguarda tutti, perché il modello europeo deve funzionare in quanto tale, la sua ragion d'essere deve esistere prima delle battaglie politiche sui contenuti: e questo non è ancora un dato pacificamente acquisito. La mia ultima considerazione ci porta più vicini alla situazione italiana ed è che il tema Europa è quello politicamente e programmaticamente più pregnante per misurare la capacità di una politica delle «larghe intese» di far fronte alle difficili sfide che abbiamo davanti. Su questo tema abbiamo misurato in passato, tra le forze che oggi sostengono il Governo, distanze culturalmente e qualitativamente significative, forse più che su altri temi. Esse possono sembrare in via di superamento, con il comune giudizio sull'inadeguatezza della politica di austerità così come si è esplicata in Europa. da più parti leggiamo oggi citazioni positive delle idee di Paul Krugman, dopo che per anni si è irriso ad ogni teoria che non discendesse dal pensiero unico della Scuola di Chicago. Ma la giusta critica ai limiti dell'austerità a senso unico non definisce da sola una politica, non delinea un orizzonte strategico, non fa da sola alleanza in Europa. può portare, ad esempio, ad assumere seriamente il tema del rigore e del risanamento, pur *cum grano salis* o con la schiena dritta, o invece a relativizzarne il valore, lasciando capire che le cose non sono così gravi e che si può sfuggire al principio di realtà. Può sollecitare nuove politiche pubbliche, intelligenti e non invasive, o invece propugnare nuove *deregulation*, nuovi conflitti tra Stato e mercato. Può rivendicare un più forte e ambizioso bilancio dell'Unione europea, che sposti al livello comunitario i grandi quadri degli investimenti, o invece chiedere di ridurlo e dare come percorribile la rinazionalizzazione di pezzi importanti della politica. Può suggerire la costruzione di relazioni nuove, dialettiche ma feconde, tra Italia, Germania, Francia, o invece proporre bracci di ferro diplomatici con la cancelliera Merkel o con la Commissione. Può infine condurci a sfidare vecchi e nuovi populismi, che si alimentano proprio delle difficoltà dell'Europa, o invece lisciare loro il pelo, visto che tra un anno si vota per il Parlamento europeo. Tra queste concezioni diverse si gioca la vera partita politica oggi. Essa va condotta seriamente sui piano valoriale, culturale e politico, a mio avviso in due modi: sul terreno delle idee e dei programmi, con il pieno e legittimo dispiegarsi dell'autonomia e dell'iniziativa di ogni forza politica; e dentro il Governo, trovando le sintesi via via più dinamiche ed efficaci, cose che oggi ritroviamo nella proposta di il Partito Democratico farà la sua parte, non nasconderemo le diversità, presenteremo il nostro disegno complessivo, ma opereremo in modo costruttivo e attivo perché il Governo e le sue sintesi politiche possano produrre buoni risultati, per l'Italia e per l'Europa tutta. Grazie, presidente Letta, per il suo lavoro.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 e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni. Passiamo quindi alla votazione della proposta di risoluzione... BARANI

Dichiaro aperta la votazione.

in uno stesso nucleo familiare convive una persona portatrice di *handicap* che chiede in questo caso al Comune di poter essere inserita in una casa di cura, e non ha alcun sostegno da parte della famiglia, nonostante i familiari, in questo caso i congiunti più stretti ovvero il fratello, godano di un reddito decisamente elevato.

Tuttavia, il percorso non è ancora concluso e non lo sarà fino a quando non sarà portato all'attenzione delle Aule del Parlamento, per poter quindi rivedere questi indici e consentire che nelle determinazioni dell'ISEE siano considerati anche in questo caso ascendenti, discendenti o parenti congiunti. Si tratta di un aspetto non semplicemente formale, per riconoscere alle persone che ne hanno bisogno il diritto di poter godere di servizi senza che altri se ne approfittino, a loro svantaggio.

per portare alla sua attenzione e a quella dei colleghi un avvenimento che rappresenta una sconfitta per la società civile e per la lotta alla criminalità. In un territorio che da anni è segnato dalla forte presenza di organizzazioni criminali, come quello compreso tra i Comuni di Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa e Casapesenna, in provincia di Caserta, la presenza di un nucleo operativo delle Forze dell'ordine rappresenta un autentico baluardo nell'ambito di una seria strategia di lotta al potere camorristico. Per effetto di apposito decreto, datato 24 maggio 1996, «al fine di rendere più efficace la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'agro aversano», veniva istituito il posto fisso operativo della Polizia di Stato di Casapesenna, alle dipendenze della questura di Caserta. Nel corso degli anni, il personale del posto fisso operativo della Polizia di Stato di Casapesenna, operante su un territorio ad altissima densità criminale, ha dimostrato, numeri alla mano, alta professionalità sia nella prevenzione che nel vero e proprio contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, all'abusivismo edilizio, al traffico di armi e munizioni da guerra e a tutte le attività che negli anni hanno inondato le casse dei potenti *clan* camorristici guidati da figure a noi tutti note, come Francesco Schiavone, Michele Zagaria, Antonio Iovine. Le 24 unità, di cui un solo ispettore, in servizio presso il posto fisso operativo hanno ricevuto ampi riconoscimenti per il lavoro svolto, lavoro che hanno messo a disposizione degli inquirenti, in quanto conoscitori esperti del territorio e del tessuto sociale su cui spesso si stende quella fitta rete criminale capace di sfuggire anche ai controlli di altre istituzioni di polizia. Purtroppo però, proprio in queste ore, per effetto dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica disposti dal Governo Monti, il Ministero dell'interno, con decreto datato 3 giugno 2013, ha ordinato la chiusura del suddetto posto fisso operativo di Polizia di Casapesenna per motivazioni legate, si legge nella bozza «all'esigenza di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, in termini di economicità, efficienza ed efficacia, mantenendo inalterata la capacità operativa della Polizia di Stato sul territorio interessato». La decisione di chiudere il posto di Polizia ha suscitato una protesta molto forte da parte della cittadinanza, che si è immediatamente adoperata organizzando una petizione sottoscritta da migliaia di persone, in quanto tale decisione rappresenterebbe la perdita dell'unico presidio di legalità in questo Comune che cerca con tutte le forze di combattere la criminalità organizzata. Lo stesso magistrato della DDA di Napoli Catello Maresca,

Pietro Grasso: un secolo di storia per un'avventura iniziata nel 1923 dal CNR, che alla sua fondazione ebbe come primo presidente il famoso matematico Vito Volterra, che ricordo perché nasce dalla sua idea. Per quanto ci riguarda, anche oggi il presidente Letta ci ha raccontato e ci ha convinto ancora una volta di quanto lo sviluppo sia importante e di quanto sia utile la ricerca scientifica nel nostro Paese e all'interno dell'Europa. Il CNR celebrerà durante l'anno questo suo novantesimo anniversario con un programma di iniziative che coniugheranno ricerca scientifica, innovazione, rapporto con i territori e soprattutto con il mondo dell'imprenditoria e della pubblica amministrazione, rinnovando quelle che sono da sempre le linee guida del CNR ispirate ai principi di autonomia, interdisciplinarità e internazionalità. Si tratta, pertanto, di un'occasione irrinunciabile per aprire un momento di riflessione e di confronto sui valori della ricerca scientifica, sulla sua importanza per la vita economica e sociale. Non dobbiamo mai considerare l'investimento nella ricerca una spesa, ma semplicemente un modo per sviluppare il nostro Paese all'interno dell'Europa. La ricerca italiana è di qualità elevata, elevatissima; troppi giovani ancora se ne vanno all'estero (il che va bene), però non ritornano perché le nostre condizioni non sono competitive per un giovane o per una persona che vuole dedicare la sua vita alla ricerca; quindi, abbiamo molto da fare. Oggi il presidente del CNR Nicolais ha ricordato quanto il CNR abbia sostenuto e favorito l'ammodernamento, la creatività, la crescita sociale e culturale, la competitività e la produttività del Paese in questi novant'anni, insieme al dialogo con imprese, istituzioni e comunità scientifiche. Pertanto, come il Ministro oggi ha ripetuto,

Grazie, presidente dal collega senatore Barani, in merito al terremoto verificatosi in Lunigiana. Collegandosi al recentissimo evento sismico verificatosi in Toscana, il collega ha testualmente detto: «Sono sicuro che la procura di Massa non aprirà fascicoli contro la scienza, come è accaduto all'Aquila, non si condannerà chi non ha previsto i terremoti, perché certe sentenze non vanno rispettate, come quella dell'Aquila, dove i più grandi scienziati sono stati accusati di non aver saputo prevenire i terremoti, facendo un danno di immagine all'Italia incommensurabile». Chiedo scusa, ma ritengo veramente gravi e inaccettabili tali affermazioni del senatore Barani. La magistratura e le sue sentenze vanno rispettate, cari colleghi, e senatore Barani, che mi spiace sia uscito. La procura dell'Aquila, nel motivare la sentenza di condanna dei componenti della Commissione grandi rischi, afferma che gli stessi componenti avrebbero dovuto «valutare il rischio sulla base delle loro effettive conoscenze e calibrare una corretta informazione». In pratica, la procura ha contestato loro una non idonea valutazione del rischio e una non idonea informazione. È stato riconosciuto da altri vulcanologi, in sede di processo, che giorni prima del terremoto c'erano parametri geofisici che facevano pensare che lo sciame stesse evolvendo, segno concreto del fatto che scienziati e tecnici si aspettavano un'evoluzione concreta del fenomeno. Insomma, il rischio c'era, eccome, e la popolazione andava informata, non disinformata. Erano stati chiamati per informare; non l'hanno fatto: il ruolo degli scienziati è stato di tipo politico, e non di carattere scientifico, nell'attività di distensione e rasserenamento della popolazione, al punto che i cittadini, nonostante la scossa di magnitudo 5.2, delle ore 23,45, si sono messi a dormire, somministrando addirittura camomilla ai propri figli, come testimoniano temi scritti dai miei alunni, che ho consegnato agli avvocati impegnati nell'inchiesta. La sentenza non c'entra nulla con la previsione *tout court* dei terremoti. Le vittime sono state dei martiri di una società che non tutela, permettendo invece alla politica di inserirsi in ruoli che non le competono

Presidente, colleghi rimasti *(Ilarità)*, il Presidente del Consiglio oggi, illustrandoci il programma che presenterà al Consiglio europeo, ha sottolineato, tra i punti salienti, la definizione di misure per favorire competitività, occupazione e crescita. Credo che possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che occorra in tutti i modi attendiamo con ansia l'inizio dell'*iter* parlamentare dei decreti cosiddetti «del fare» e «semplificazione». gli interventi cui provvedere al più presto, perché a costo zero, capaci di creare risparmio e di rapida e agevole fattibilità, figura sicuramente l'abbattimento degli ostacoli burocratici, che congelano l'iniziativa privata e l'economia e rallentano la nostra uscita dalla crisi che ci sta tormentando. Al riguardo, molti i casi di facile soluzione, e sicuramente il mio Gruppo, già intervenuto in merito con alcuni emendamenti del DEF, continuerà fattivamente a dare il suo supporto quando sarà il momento. Oggi, considerando le mie competenze specifiche, nonché l'incombenza di un obbligo burocratico a scadenza molto prossima, ovvero il 30 giugno, vorrei sottoporre alla vostra attenzione un obbligo che incombe come una spada di Damocle su molti medici competenti e che si palesa in un esempio emblematico dell'inutilità di alcuni vincoli burocratici, mal concepiti e condotti, che si traducono di fatto in un freno nel mondo del lavoro e in un ostacolo a percorsi più virtuosi. Sto parlando dell'articolo 40, e del relativo allegato 3B, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Il Governo ha inteso apportare modifiche volte alla semplificazione anche in materia di lavoro, specialmente finalizzate a rimuovere obblighi di natura esclusivamente formale con scarsa rilevanza in termini di effettivo risultato sui livelli di tutela della Le semplificazioni riguardano principalmente gli obblighi aziendali relativi alle figure del datore di lavoro, dei dirigenti e in alcuni casi anche del RSPP, del rappresentante degli stessi lavoratori, ma incomprensibilmente non è stata presa in considerazione la figura del medico competente, titolare di compiti e obblighi fondamentali per la tutela della salute dei lavoratori, cui peraltro la legge attribuisce attualmente anche oneri burocratici caratterizzati da estrema difficoltà applicativa e di dubbia validità ed efficacia in termini di risultato, come l'obbligo previsto dall'articolo 40 e relativo allegato 3B del

ad oggi il SINP, Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e premessa necessaria ai fini di una razionale e fruibile raccolta di dati epidemiologici, non è ancora attivo. Per